è legittimo e non può essere legittimato - e la politica dovrebbe dire parole chiare su questo - è che dei manifestanti vadano sotto casa di cittadini o dello stesso amministratore della città, perché ciò diventa pericoloso

quindi davvero esprimere, a nome di tutto il Gruppo dei senatori del Partito Democratico, solidarietà al sindaco di Pesaro e a tutti i sindaci che si trovano ad affrontare particolari situazioni, sperando di poter condividere questo momento con tutti i colleghi dell'Assemblea.

Viva-PSI, vicinanza e amicizia al sindaco Matteo Ricci e ai tanti amministratori che si stanno trovando nelle stesse difficoltà. Come diceva la collega Malpezzi, infatti, le manifestazioni, quando autorizzate, sono sempre legittime; quando invece si arriva a questi livelli e si supera evidentemente il limite della manifestazione normale e autorizzata, allora è giusto anche anche far comprendere ai tanti cittadini, che in questo momento magari sono arrabbiati e preoccupati, le ragioni di scelte sicuramente difficili, ma coraggiose e di grande responsabilità,

n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, prevede una serie di misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia. Il provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia riunite, che hanno apportato modifiche puntuali al testo, anche con la collaborazione dell'opposizione, che ovviamente ringraziamo. Da parte delle forze politiche c'è stata, anzitutto, la consapevolezza dell'importanza di un provvedimento che affronta il reclutamento come lo strumento grazie al quale i progetti previsti dal PNRR saranno messi a terra dalle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali. Per fare questo, è stato chiaro a tutti, sin dal primo momento, che servono risorse, capacità e talenti specializzati e motivati, ma che serve anche individuare procedure adeguate. Questo decreto lo fa in maniera equilibrata, tenendo conto degli interessi in campo e delle garanzie necessarie. Per il lavoro fatto, permettetemi di ringraziare in modo particolare la sottosegretaria Bini, il ministro D'Incà, il Governo in generale e, ovviamente, il Ministro per la funzione pubblica e la Ministra della giustizia, direttamente interessati, così come tutti i loro uffici. Ringrazio poi tutti i colleghi della Commissione affari costituzionali e della Commissione giustizia, così come tutti i funzionari e il personale del Senato. Per limiti di tempo, darò conto in particolare solo di alcune modifiche intervenute in sede parlamentare nel lavoro delle Commissioni. Per quanto riguarda il rafforzamento della capacità amministrativa, l'articolo 1 disciplina modalità speciali per accelerare le procedure per il reclutamento di personale a tempo determinato e il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel PNRR. Per quanto riguarda gli elenchi introdotti all'articolo 1 del decreto, istituiti attraverso il portale del reclutamento dal Dipartimento della funzione pubblica per accelerare le procedure concorsuali, è stata introdotta una modifica, che prevede l'estensione dell'iscrizione anche a quei professionisti non organizzati in ordini e collegi in possesso dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi. Inoltre, tutti i bandi sul portale del reclutamento saranno pubblicati in formato aperto e organizzati in un *database* ricercabile in ogni campo. È stato poi prorogato al 31 dicembre 2022 il termine entro cui le amministrazioni, per superare il precariato, possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale secondo i termini di legge già stabiliti. Sono state previste misure urgenti legate all'attuazione del PNRR che riguardano il Ministero della cultura, con l'assunzione di personale specializzato destinato agli archivi di Stato e alle sovrintendenze archivistiche. Andando all'articolo 3 - che interessa la disciplina concernente l'inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali, la progressione all'interno dell'area e l'accesso ad aree superiori - una serie di modifiche introdotte in Commissione hanno riguardato, in particolare, le progressioni nella stessa area, che debbono avvenire secondo principi di selettività e in funzione delle capacità maturate secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. È stato inoltre previsto che nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, Regioni ed enti locali a tutti i soggetti con DSA sia garantita la possibilità di sostituire le prove con un colloquio orale, usando strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo. Sul tema della mobilità volontaria, tanto sentito tra le pubbliche amministrazioni, il decreto interviene limitando i casi in cui essa è subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Su questo, recependo i dubbi sollevati dagli enti locali, è stata trovata una soluzione soddisfacente, mantenendo il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nei Comuni fino a 100 dipendenti e riducendo la percentuale corrispondente alla carenza di organico che lo renda necessario. Inoltre, per tutti gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale diventa di cinque anni. Sempre per gli enti locali, è stata introdotta un'innovativa modalità aggregata tra di essi per la gestione delle selezioni, in vista degli elenchi di idonei all'assunzione, a tempo sia determinato sia indeterminato. All'articolo 4 del decreto, che concerne le funzioni e la struttura dell'associazione Formez PA, è stata introdotta in Commissione una modifica sulla composizione del Consiglio di amministrazione dell'associazione, dove i membri in rappresentanza di Regioni, Unione Province d'Italia Nel testo del decreto è stato poi inserito, come emendamento presentato al Governo, il decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica (Mite) e in materia di sport. Le principali disposizioni sono rivolte all'assunzione di personale specializzato presso il Ministero della transizione ecologica. poi in materia di struttura di missione per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Mite. È prevista, infine, la nomina da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro della transizione ecologica di un inviato speciale per il cambiamento climatico, con il compito di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali. Oltre ad alcune disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), si interviene sullo scopo statutario della società pubblica *Infrastrutture Milano Cortina* 2020-2026 SpA. Infine, in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpionico nazionale italiano (CONI), si rimanda allo stesso la facoltà di definire l'articolazione della propria dotazione organica, nonché i criteri e le modalità per il reclutamento del personale finalizzato al completamento della medesima. L'articolo L'articolo 6 del decreto introduce per le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti un Piano integrato di attività e organizzazione che riguarda, tra gli altri, i profili legati a *performance*, capitale umano, organizzazione, trasparenza e anticorruzione. In Commissione, il termine per presentare il Piano è stato fissato al 31 gennaio di ogni anno, inserendo anche l'obbligo di assicurare adeguata informazione alle organizzazioni sindacali. Si è previsto inoltre che gli enti locali con meno di 15.000 abitanti possano provvedere al monitoraggio previsto dal Piano individuando un ufficio associato a livello provinciale o metropolitano. Sempre all'articolo 6, comma 2, gli strumenti definiti dal Piano per raggiungere gli obiettivi in materia di trasparenza e anticorruzione saranno definiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e agli indirizzi dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), con l'obiettivo, da un lato, di salvaguardare l'intento semplificatore all'origine del piano e, al contempo, di armonizzare questa disciplina con le funzioni in capo all'autorità anticorruzione. All'articolo 9 del decreto-legge le risorse previste per gli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che gli enti territoriali attiveranno per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del Piano sono state aumentate per ciascuno degli anni 2021-2024. Per quanto riguarda la giustizia amministrativa, si è intervenuto con alcune norme per facilitare lo svolgimento dei concorsi già previsti dal provvedimento, inserendo come titolo di preferenza, a parità di merito, anche il diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali. Altre norme inserite in Commissione riguardano l'attuazione in ambito di giustizia amministrativa del Piano di ripresa e resilienza e l'incentivazione per favorire la partecipazione dei magistrati al piano di smaltimento. Vorrei infine ricordare che la Commissione ha voluto inserire all'articolo 17 quello di parità genere come principio guida anche per il piano di reclutamento del personale a tempo determinato previsto dal decreto-legge. ne restano ancora aperte altre. Ne indico due note all'Assemblea, riguardanti alcuni nodi sulla giustizia e in modo particolare alcuni legati a quella amministrativa, che meriterebbero di essere affrontati superando lo spirito corporativo e guardando invece alla funzionalità dell'amministrazione della giustizia. Mi auguro che il lavoro prodotto su entrambi i fronti durante queste settimane non venga abbandonato e possa essere ripreso al più presto in una prossima occasione.

positiva. Durante il lavoro in Commissione, abbiamo introdotto alcune correzioni, che devono determinare una maggiore capacità di intervento. In particolare, si è tolto l'obbligo del rapporto del rapporto da remoto effettuato tra i nuovi, laureati in legge o in economia, che devono collaborare con il giudice. Dipenderà molto dai coordinatori dei vari uffici del processo, nelle varie zone d'Italia, attivare un rapporto diretto tra giudice e collaboratori. Basta leggere il primo profilo di quello che saranno chiamati a svolgere: oltre ad alcune attività più semplici, come la verifica della correttezza del fascicolo processuale, hanno anche la possibilità di collaborare con il giudice nel predisporre bozze di provvedimenti

possa intervenire tenendo conto di quanto ha detto la Corte costituzionale negli ultimi tempi in merito alla magistratura onoraria. Colleghi, consentitemi alcune

La vera attività in Parlamento è quando forze politiche diverse si incontrano per realizzare un prodotto che abbia una sua effettività. Faccio un esempio:

Rispetto a questa situazione, dobbiamo assumere una responsabilità, che per gran parte siamo riusciti a prenderci, ma forse dobbiamo fare uno sforzo ulteriore,

abbiamo accolto come relatori e come Governo. Questa logica di collaborazione tra Governo e Parlamento può muoversi soltanto su una linea, e lo dico anche

che le correzioni introdotte con lo spirito a cui ho fatto cenno possano eventualmente essere integrate anche in questa sede oppure essere condivise, ma nella realtà. Infatti, la norma, una volta licenziata dal Parlamento, assume una sua realtà completamente diversa, che è rimessa all'interprete, ma anche alla capacità dei dipendenti, di coloro che svolgono la propria attività nella pubblica amministrazione e dell'amministrazione della giustizia di attuare in concreto i singoli provvedimenti.

nella sua lucidità di pensiero, che gli voglio riconoscere in questa sede e che, almeno per me, rappresentano una guida anche per il mio futuro politico.

il suo modo di lavorare, la sua disponibilità verso gli altri e la sua incredibile pazienza, fino al punto che l'altra sera ha detto di non sentirsi bene, perché si era molto stressata, ma il giorno dopo l'ho vista di nuovo al lavoro. Quindi complimenti e congratulazioni - se li merita - al

di forte confronto, ma la politica è questo ed è bella per questo: anche da posizioni differenti, ci si confronta e si deve avere la capacità di raggiungere una sintesi. Devo dire che questa è stata una di quelle occasioni nelle quali anche posizioni di partenza molto differenti hanno trovato un loro momento di sintesi.

Siamo fatti così: siamo un partito liberale e ci definiamo un partito del fare, che, come ha ricordato poco fa il collega Caliendo, non vuole mettersi delle stellette per dire che qualcosa l'abbiamo fatto noi,

su molti altri si sono astenuti, anziché votare contro. Credo che questo sia lo spirito giusto per affrontare un momento del Paese particolarmente difficile. L'ho detto, lo ripeto e lo ripeterò ancora: la classe dirigente di questo Paese deve saper dimostrare in questo momento grande carattere e grande senso di responsabilità, e non è un modo di dire, perché è fondamentale. Al futuro degli italiani ci dobbiamo pensare oggi, adesso, perché le decisioni che stiamo assumendo in queste ore, in questi giorni, varranno per i prossimi anni per il nostro Paese. Se pensiamo che l'indice di crescita già prima del Covid era molto basso e poi, durante il periodo della pandemia, è crollato, come in altri Paesi in tutto il mondo, dobbiamo essere consapevoli che con questo Governo abbiamo la possibilità di raggiungere indici di crescita non

stiamo cercando di migliorare anche in sede parlamentare. Egli, quindi, avvia il processo e noi parlamentari abbiamo il dovere di migliorare le sue indicazioni. Tutti noi anche in questa circostanza, così com'è stato

fa sì che il Gruppo Forza Italia rappresenti davvero un punto di riferimento fondamentale non solo per il *Premier* e per il Capo dello Stato, ma per il popolo intero.

che dovrebbe rappresentare il raggiungimento di un obiettivo che per noi è sempre stato quasi una chimera, cioè la spesa dei fondi che ci verranno dati.

avanti ed avere, cari colleghi, la capacità di cambiare, di modificare il nostro modo di fare, di realizzare quella spesa che non abbiamo potuto fare. Lo facciamo attraverso

ma che ringrazio - che ha avuto insieme a me e ad altri colleghi eletti nella Regione Abruzzo, la capacità di mettere in risalto e di coinvolgere tutte le forze politiche, nessuna esclusa, anche quelle

che non dovevano chiudere, con questo provvedimento e con l'aiuto di tutte le formazioni politiche abbiamo combattuto tutti quanti insieme e abbiamo dato una bella dimostrazione di coesione e di capacità di venire incontro alle esigenze del territorio per un miglior funzionamento ed efficientamento del sistema della giustizia, in questo caso in Abruzzo e in futuro mi auguro con una diversa geografia Grazie a tutti e buon lavoro.

il nuovo percorso della pubblica amministrazione, con il progressivo abbandono del modello burocratico in favore di un approccio aziendalistico, ha origini ormai risalenti nel nostro impianto legislativo. La vecchia struttura organizzativa gerarchica, seppur con difficoltà, è stata via via sostituita da un approccio manageriale e da una nuova visione del lavoro non più ancorata al concetto di mansione, ma organizzata per il raggiungimento di obiettivi secondo una logica di risultato. L'urgenza di garantire un modello di gestione efficace e un'adeguata disponibilità di competenze si affianca all'esigenza di ringiovanire la pubblica amministrazione e di garantire un organico efficiente. La pandemia e tutte le difficoltà che ne sono derivate hanno reso ancora più evidenti i problemi presenti nella nostra pubblica amministrazione. Le carenze di organico specializzato, la scarsa valorizzazione delle competenze e soprattutto un'età media dei dipendenti troppo alta, che si attesta intorno ai cinquant'anni: sono queste alcune tra le storture che è necessario risolvere. La necessità, quindi, di rendere attrattiva la pubblica amministrazione per convogliare al suo interno risorse umane e competenze di eccellenza trova nel PNRR nuova linfa vitale, aprendo una stagione di investimenti pubblici e di auspicata rinascita. Dopo anni di tagli e di *austerity*, finalmente ritroviamo risorse e ossigeno per le riforme, per poter così scommettere sul capitale umano, per investire nella valorizzazione del merito e per attrarre giovani professionisti. Il decreto che ci apprestiamo a convertire si inserisce in questo solco. I suoi 19 articoli puntano puntano tutto sul capitale umano, istituendo percorsi semplificati e straordinari per rafforzare la capacità amministrativa della pubblica amministrazione e della giustizia, prevedendo percorsi trasparenti, veloci e definiti. Il titolo I si apre con la previsione di modalità speciali per conferire incarichi professionali dando la possibilità alla pubblica amministrazione di porre a carico del PNRR solo le spese per il reclutamento del personale destinato a realizzare i progetti di cui le singole amministrazioni hanno titolarità diretta di attrazione, prevedendo la possibilità di ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato e a contratti di collaborazione anche per un periodo superiore a trentasei mesi, con il solo limite temporale posto al 31 dicembre 2026. Tali contratti dovranno indicare il progetto del PNRR cui saranno riferiti, potranno essere rinnovati e prorogati per una sola volta e saranno sottoposti a valutazione di risultato. Al fine di non sprecare le competenze maturate, valorizzare l'esperienza e consolidare le capacità, sarà possibile riservare una quota di posti, non superiore al 40 per cento, nei bandi dei concorsi successivi per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, in favore del personale reclutato ai fini dell'attuazione del PNRR che, al momento della pubblicazione del bando, abbia maturato un'esperienza di almeno trentasei mesi all'interno

di carriera. Inoltre, l'emendamento interviene sulla valutazione delle esperienze maturate, dando peso alla tipologia e non al numero degli incarichi, nella convinzione che sia preferibile un criterio qualitativo rispetto ad un criterio quantitativo. Per quanto riguarda il settore giustizia, il decreto fissa nuove misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa, al fine di favorire l'operatività dell'ufficio per il processo e di assicurare lo smaltimento dei procedimenti giudiziari arretrati. Il Ministero della giustizia potrà avvalersi delle piattaforme digitali della pubblica amministrazione per avviare procedure di assunzione per 16.500 unità con contratti di lavoro a tempo determinato e di 326 unità per la giustizia amministrativa. Il servizio svolto con merito dai soggetti in possesso di laurea in giurisprudenza potrà valere come titolo per accedere al concorso in magistratura ordinaria, ovvero come tirocinio professionale per l'accesso all'esame di Stato da avvocato o al concorso concorso notarile. Sarà poi il Ministro della giustizia a individuare tribunali e corti di appello cui destinare le risorse, nonché il numero degli addetti per ogni singolo ufficio. Sarà possibile, inoltre, per il Ministero della giustizia avviare procedure di reclutamento tramite concorsi per titoli o prova scritta. È poi espressamente previsto il criterio dello scorrimento delle graduatorie, anche per diverse tipologie di concorsi per diversi distretti giudiziari, laddove una graduatoria risultasse incapiente. Il personale così reclutato sarà impiegato per lo smaltimento dell'arretrato, preferibilmente in modalità da remoto, anche nell'ottica della transizione digitale, Grazie a tutti

Grazie

soprattutto in coloro che hanno avuto la fortuna, oltre che l'onere, di essere amministratori e di conoscere le vere condizioni nelle quali versa l'amministrazione pubblica in Italia, sapendo quanto è difficile mietere un risultato, in particolare quando si è al cospetto di un ambizioso lavoro che, come veniva detto, ricadrà sulla vita della nostra Nazione nei nei prossimi anni. Quando si tratta di rafforzare il capitale umano della pubblica amministrazione, magari elevando anche la qualità professionale e abbassando il dato anagrafico, per noi di Fratelli d'Italia si tratta sempre di un momento importante, anche se dobbiamo dire che

che, dopo anni di blocco del *turnover* e di mancate assunzioni, la nostra amministrazione pubblica era incapace di era incapace di gestire anche l'ordinaria amministrazione, con una ricaduta negativa in termini di servizi da dare ai cittadini, alle imprese e a tutto quel tessuto sociale che opera nei territori e che naturalmente si aspetta ben altre risposte in termini di efficienza e di velocità. di velocità. Come ho detto in altri interventi, da amministratore locale ho conosciuto anche storie straordinarie di professionisti che hanno fatto la scelta della

più lauti di quelli che ricevono dallo Stato. Essi hanno invece scelto di servire la missione pubblica e a loro vanno

che anche in questa occasione dimostrano tutta la loro fragilità. La maggioranza ci sembra infatti un gigante dai piedi d'argilla, soprattutto se ci troveremo al cospetto dell'ennesimo voto di fiducia. io voglio ringraziare il sottosegretario Bini, per la cortesia dimostrata nelle occasioni di confronto politico, la prima cosa che abbiamo chiesto, visto il nostro atteggiamento assolutamente aperto, collaborativo e costruttivo nell'interesse della Nazione, era che non venisse posta la questione di fiducia. Ci sembra però che ci si avvii a questo, dopo il pomeriggio

amministrazione, ci sono alcune vicende politiche che spero che già il Consiglio dei ministri di questa mattina voglia affrontare, perché rappresentano una vera e propria emergenza. Signor Sottosegretario, non conosciamo ancora la data delle elezioni amministrative. È possibile che nell'unica Nazione in Europa in cui le elezioni sono state rinviate, nell'unica Nazione in Europa in cui le elezioni sono state rinviate, non si conosca ancora la data delle elezioni amministrative? Abbiamo sindaci sostanzialmente in proroga dobbiamo mettere in piedi tutta l'architettura politica e partitica delle liste, ma ancora non conosciamo la data delle elezioni.

è materialmente impossibile e se non vogliamo che oltre 10 milioni di cittadini italiani vivano in Comuni falliti,

rafforzare la capacità amministrativa del sistema e sopperire alla carenza di professionalità tecniche diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa; potenziare le infrastrutture digitali; garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne. Partendo da questo presupposto,

anche la possibilità di investire sulle risorse umane, che, come ho detto prima e anche in altre occasioni, rappresentano la vera e propria benzina da immettere all'interno di un motore che, purtroppo, è stato abbandonato.

Grazie a tutti

ma potremmo prendere ad esempio molti altri tribunali, che lavorano solo perché ci sono delle persone che vanno al di là dei loro limiti e di questo li dobbiamo ringraziare. All'interno di questo provvedimento si va ad incidere Sicuramente è positivo il fatto che noi oggi ci prendiamo un impegno nei confronti della macchina della giustizia e nei confronti dei cittadini. Ci prendiamo un impegno, che ovviamente poi il Governo e noi tutti in Parlamento dobbiamo portare a piena attuazione.

Grazie a tutti

obiettivamente è stato creato per cercare di risolvere un problema, ma probabilmente ne crea degli altri, quantomeno all'interno della gestione della macchina amministrativa e della macchina giustizia. vive il tribunale, perché chi non ha modo di lavorare all'interno delle stanze dei tribunali, probabilmente non sa nemmeno che cos'è l'ufficio per il processo. Poi, nel concreto,

che, all'interno di tutte le riforme che stiamo portando avanti, a cominciare da questa, dobbiamo cercare di immettere quelle risorse di cui parlavo prima,

qualcosa di positivo in una macchina che però sta ferma. Non dobbiamo permettere questo, ma dobbiamo consentire invece che la macchina corra, nel rispetto del diritto, all'interno di tutte le altre rivoluzioni che stiamo vedendo, come la riforma del processo civile e del processo penale, stiamo guardando sempre e soltanto a quello che ci dice l'Europa all'interno delle indicazioni del Piano, cioè che la giustizia deve essere veloce. Aggiungo che la giustizia deve essere veloce, ma deve essere giusta, deve essere giusta, nel rispetto delle norme di diritto dell'ordinamento giudiziario e dell'ordinamento giuridico, altrimenti veniamo meno a quei richiami che sono all'interno della Costituzione e che dobbiamo continuamente tenere a mente, tutti noi che lavoriamo all'interno delle Aule legislative.

Parlamento, però dobbiamo ricordarci che quando parliamo di rafforzamento della pubblica amministrazione e rafforzamento della giustizia, dobbiamo farlo due elementi: rapidità e oculatezza. Qui mi rivolgo al Sottosegretario, che ringrazio per la pazienza che ha avuto durante le sessioni di Commissione, a tratti estenuanti, ma, obiettivamente, io credo che si poteva

sprecate. Non voglio dilungarmi oltre, ma ricordo semplicemente che la riforma della giustizia, la riforma del personale della giustizia e di tutti coloro che lavorano all'interno della giustizia non si ferma al 2026. Noi dobbiamo lavorare oggi, affinché tutto il sistema giustizia vada a regime e vada a regime seriamente. Su questo faccio un ultimo richiamo, ricordando il monito che il presidente dell'Unione camere civili ha fatto all'ultimo Congresso nazionale forense, in cui ha detto, molto chiaramente, che non bisogna dimenticare che la giustizia giusta non sempre è giustizia veloce e viceversa. Quindi, noi lavoriamo affinché sia il più veloce possibile, ma sempre nel rispetto dei diritti dei cittadini. cittadini. Mi rimetto alle dichiarazioni di voto del mio Gruppo. Ringrazio dell'attenzione e, ovviamente, mi auguro che i provvedimenti arrivino realmente nelle aule dei tribunali e nelle aule della pubblica amministrazione, affinché tutti i cittadini possano avere finalmente un servizio quantomeno

della pubblica amministrazione, consentitemi di fare una riflessione sul mio percorso professionale. Io sono stata venticinque anni nella pubblica amministrazione. La sensazione che ho sempre avuto è stata che la forma e il rigore procedurale fossero molto più importanti della sostanza e degli obiettivi, che le relazioni con il mondo politico fossero molto più importanti dell'apporto professionale individuale, magari talvolta critico, e che il lavoro individuale fosse più importante di quello in *team*. Concludo dicendo che anche la comunicazione, se troppo chiara e trasparente, veniva considerata meno professionale rispetto al cosiddetto linguaggio burocratico. Poi sono passata a lavorare nel privato e mi sono resa conto che la situazione era esattamente contraria. Quindi, mi sono chiesta perché alcune funzioni, più tipiche del mondo privato, non entrassero nella pubblica amministrazione e il cosiddetto rigore procedurale, più tipico della pubblica amministrazione, non permeasse invece il mercato. Dico questo perché, secondo me, è fuorviante pensare che vi sia una contrapposizione tra mercato e pubblica amministrazione, che invece devono poter coesistere in maniera equilibrata e complementare. Un'economia sana è sicuramente un'economia che ha bisogno di entrambi gli aspetti: di buone regole, di servizi pubblici di qualità e di imprese dinamiche ed innovative. Ricordo, peraltro, che il *premier* Draghi ha detto che il *recovery plan* può, ma soprattutto deve, essere un grande attivatore di investimenti privati, una sorta di leva finanziaria per sollevare l'economia del Paese. Queste sono parole che hanno un peso specifico estremamente importante. Io credo che tutti noi siamo oramai convinti, perché lo stiamo dicendo nei lavori di Commissione, in Aula e dappertutto, che il *recovery plan* offra la possibilità di migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione, di stimolare l'iniziativa privata e quindi di modernizzare l'economia. Senza alcuna enfasi eccessiva, ma con assoluto pragmatismo, visto che la politica deve essere anche pragmatica e non solo dogmatica, possiamo dire che dal successo delle riforme, dagli interventi, dai progetti di ampio respiro del *recovery dipenderanno le opportunità che l'Italia offrirà alle prossime generazioni. La parola riforme ricorre moltissimo; consentitemi allora una riflessione sul riformismo moderno. Ne ho sentito parlare la prima volta che mi avvicinai alla politica, nel lontano 1989. Non mi riferisco al riformismo *tout court*, ma al riformismo socialista per richiamare quella attitudine

da un lato, e alla filosofia - lasciatemela passare così - del tirare a campare di stampo democristiano, dall'altro. Sto parlando quindi di una vocazione al cambiamento e soprattutto della modernizzazione del nostro Paese. Come si fa la modernizzazione di un Paese? Con un atteggiamento mentale di ottimismo della volontà con il quale si deve assolutamente guardare al futuro. Se io oggi dovessi, alla mia età, ritornare a lavorare nella pubblica amministrazione, cavalcherei veramente la voglia di cambiamento e di modernità per combattere quell'immobilismo e quel conservatorismo che comunque abbiamo riscontrato ancora nei primi due decenni del nuovo secolo. Peraltro l'immobilismo e il conservatorismo sono tra i principali fattori alla base della sostanziale stagnazione economica del nostro Paese,

C'è sempre stata una dinamica molto insoddisfacente della produttività del settore dei servizi, nella quale la pubblica amministrazione ha un peso sicuramente rilevante.

la *spending review*, i centri di costo, le valutazioni delle *performance*, che peraltro sono state declinate con gli stessi parametri in tutti i settori della pubblica amministrazione, quando sappiamo perfettamente che ci sono settori

state prodotte montagne di carta, hanno funzionato. Direi di no perché se avessero funzionato, non ci ritroveremmo in questa situazione. Bisogna porsi queste domande perché analizzare i margini di miglioramento, che sono veramente tanti, è importante perché comunque le risorse spese per il

a spendere ancora di più, perché comunque si parla di assunzioni importanti, dobbiamo, indipendentemente dal parametro afferente la misura percentuale - possiamo infatti anche spendere più del 45

Sappiamo che nella pubblica amministrazione il rapporto di lavoro è di lungo periodo; si sviluppano competenze specifiche che non sono assolutamente spendibili in maniera immediata altrove, quindi, riformare i concorsi

alla quale assegnare un certo punteggio nel momento del concorso. Ancora, ho visto che i tetti di spesa relativi al trattamento economico accessorio possono essere superati. Questa è una buona notizia, il suggerimento è cercare di utilizzare le premialità per favorire il *turnover* che aiuta ad ampliare le cosiddette competenze

che funzionano - mi permetto di dire - non troppo bene. Quindi, va assolutamente ripensato il controllo esterno della Corte dei conti che, secondo me, deve essere sempre più avvicinato al modello organizzativo del Government accountability

dell'amministrazione e faccio una raccomandazione rispetto al Piano integrato di attività e organizzazione, nella speranza che non sia un *dossier* insormontabile di pagine e pagine non chiare, non trasparenti e soprattutto non produttive in termini di dati.

sentito propositi fiduciosi e molti ringraziamenti profusi a beneficio del lavoro svolto. Sinceramente il ruolo di guastafeste non mi si addice e non mi piace neanche più di tanto, in questa fase e ragionando di questo provvedimento, debbo farlo, purtroppo. Il motivo è che che noto in questo testo una sorta di buco abbastanza corposo che riguarda il complesso del sistema sanitario nazionale. Nel nazionale. Nel momento in cui si parla di riformare le procedure di reclutamento e di strutturazione del pubblico impiego,

maggiore rispondenza tra qualità del risultato e sforzo profuso per ottenerlo, anche in termini di costo. Rispetto alla

Governo - che questo provvedimento, come sapete, destina appena l'8 per cento di risorse al comparto sanità. Questo provvedimento, che non si capisce bene in quale misura agisca anche nel comparto sanità (non è chiaro e aspetteremo di vedere i decreti attuativi), semmai

ulteriormente. Nella sanità c'è bisogno di assumere. Nell'intera vicenda del Covid abbiamo assunto a tempo indeterminato poco più di 1.000 persone. Il *turnover* fino al 2020, per effetto dei pensionamenti e dei licenziamenti volontari (che sono stati tanti), ammonta

a tempo indeterminato, in sostituzione di circa 5.000 pensionamenti e circa 3.000 dimissioni volontarie. La nazionalità maggiormente

formiamo medici e professionisti straordinari, ce ne facciamo carico in termini di costo di formazione e, a causa della cecità e di una aziendalizzazione malintesa e fraintesa, questi medici e professionisti mettono il naso dentro il Servizio sanitario nazionale, sentono

qualora abbia la capacità di incidere, vedo solo ulteriore capacità di precarizzare. Eppure ci sarebbe da fare. Considerate, colleghi, che tra la decisione di assumere un medico e la sua presa in servizio in Italia ci vogliono più o meno due anni, quindi ben venga un provvedimento che snellisca queste farraginosità. Ben venga, e ci mancherebbe se noi non ne fossimo consapevoli. Ma questo non può avvenire attraverso la precarietà, perché il medico non si fa precarizzare; il medico giustamente vuole essere strutturato

che, utilizzando questo provvedimento, agiamo ulteriormente in termini di precarizzazione. E questa non è certamente la strada.

Ancora non abbiamo colmato, come ho detto poco fa, neanche lontanamente la misura necessaria, ma a questo punto dobbiamo immediatamente agire - a valle o a monte, come preferite - sull'assurdità del numero chiuso. Adesso risolveremo aumentando le borse di di specializzazione, ma se non liberiamo il tappo del numero chiuso non avremo medici professionisti disponibili a specializzarsi. Dobbiamo contrattualizzare da subito gli specializzandi al quarto e al quinto anno e lo dobbiamo fare nei servizi sanitari regionali, nella rete ospedaliera. In questo modo probabilmente, se riuscissimo a togliere di mezzo quel cattivo odore che il Servizio sanitario nazionale emana, forse riuscissimo a tenerli anche in Italia.

la nostra posizione rispetto al Governo e ai temi trattati, la nostra collocazione all'interno di questo Governo, le speranze che noi affidiamo

senatore Caliendo, il quale ci richiama sulla funzione della politica parlamentare, che abbiamo dimenticato: il Parlamento parla, discute dialetticamente, affronta le questioni

il suo discorso in un certo senso richiama Rousseau, ma lo supera. Lo dico a gli amici 5 Stelle che tanto amavano la citazione di un importante filosofo, ma il tema evidentemente lo ricolloca all'interno della funzione della politica,

la capacità di determinare i fini non appartiene alla politica, ma alla tecnica, che li sposta di volta in volta, quindi il rapporto tra mezzo, uomo e tecnica ha cambiato i nostri paradigmi. Passando al decreto-legge, la parte della giustizia va collegata evidentemente al gran lavoro che si sta facendo sulla riforma del processo civile e penale, parzialmente, ancora *in nuce*, dell'ordinamento giudiziario. Timidamente affrontiamo, nonostante il caso Palamara e tutto ciò che abbiamo visto, la riforma del Partiamo da un dato: lo smaltimento dei processi. L'Italia non sta andando male, nel senso che riusciamo a definire più processi di quanti ogni anno entrino nelle aule dei tribunali. Questo è un problema, perché vuol dire che abbiamo meno lavoro,

quattro anni, un processo civile sette anni, il collo di bottiglia lo abbiamo nel processo d'appello e nella Cassazione, guarda caso, è una tragedia. La legge Pinto stabilisce che il processo di Cassazione deve durare un anno, da noi dura anni. Venendo agli aspetti

decreto. Con spirito assolutamente collaborativo - mi piacerebbe che fosse presente il ministro Cartabia - dico che immaginavo che nella funzione dell'ufficio per il processo ci fosse la costruzione dell'ufficio per il processo del giudice costituzionale o del giudice della Corte suprema americana,

nei tribunali, nella pubblica amministrazione possiamo cambiare il volto di questo Paese e renderlo più efficiente. Abbiamo bisogno di giovani, di informatici e così

che in un grande tribunale e in una grande procura i problemi di organizzazione del lavoro siano affrontati con metodi per cui non si sa chi fa che cosa e chi decide che cosa cui la funzione del giudicante non può essere in contrasto o in collisione con quella della gestione dell'ufficio del personale e del cancelliere.

Non siete arrivati infatti nemmeno al monocameralismo. Siamo all'interno di un bicameralismo che non riesce a rappresentare i territori e le reali esigenze della gente. Sposo quindi sin d'ora l'idea di una Costituente che affianchi il sistema elettorale. La proposta della Fondazione Einaudi è giusta e ragionevole. Chiudo, infine, su una questione di attualità. Trovo fuori luogo alcune polemiche sul cosiddetto lodo prescrizione e sulla soluzione che è stata individuata dal ministro Cartabia. La vera soluzione alla prescrizione è il ritorno ad una legge che poi, in fin dei conti, non era neanche male, vale a dire la ex Cirielli *(Applausi)*: solo Cirielli si era accorto di non aver fatto una buona legge.

è l'unica soluzione possibile, anche se non è quello che vogliamo, perché parlare di improcedibilità non ha a che fare col diritto sostanziale, è questo il tema (il professor Spangher, che è stato il mio professore, lo ha ricordato in questi giorni). Se però non ci sono altre strade, dobbiamo andare lì; dobbiamo uscire da quel *monstrum* che avrete creato e riportare nei binari giusti una funzione giurisdizionale e giudiziaria che non può essere eliminata.

Signor Presidente, cari colleghi, mi concentrerò sulla parte di questo decreto-legge che riguarda il tema della giustizia, perché di competenza della Commissione di cui sono Vice Presidente. Vorrei partire dagli obiettivi che il ministro Cartabia ci ha illustrato, quando è venuto in Commissione giustizia, cioè la riduzione del 25 per cento dei tempi attuali della giustizia penale

Tutti sappiamo quanto costano alla nostra economia questo cronico ritardo e queste cronache inefficienze della giurisprudenza italiana. È un obiettivo che ci ha posto l'Europa e al quale dobbiamo assolutamente tendere, se vogliamo che, dopo i primi 25 miliardi, arrivino anche gli altri fondi del PNRR. Ebbene, qual è la risposta, qual è il programma del Governo per ottenere questo risultato? Una riforma del processo penale che, come sappiamo, è già impantanata nelle liti interne della maggioranza e una riforma del processo civile che, chi ha letto, si rende conto che è stata costruita probabilmente da teorici che vivono all'interno dei Ministeri, ma che non hanno mai messo piede in un'aula di giustizia. Insieme a queste due riforme, che purtroppo sono due riforme sprecate, per come si preannunciano,

in due scaglioni, assunti a tempo determinato: il primo scaglione per due anni e sette mesi e il secondo scaglione per due anni. E voi pensate davvero che in questo modo riusciremo a ridurre del 40 per cento i tempi della giustizia? Me lo auguro, ma temo purtroppo che non sarà così. In due anni e sette mesi, o peggio ancora in due anni, ci sarà appena il tempo di formare questi giovani, che entreranno da precari nel mondo della giustizia e che fra due anni o tra due anni e sette mesi ci dovremmo poi porre il problema di come stabilizzare. Per queste persone in molti tribunali non c'è nemmeno il posto fisico. Queste persone dentro i tribunali dovrebbero andare a coadiuvare dei giudici, che sono giustamente abituati, perché la funzione giurisdizionale è esercitata dal giudice e non dai suoi ausiliari, a esaminare il fatto, a esaminare il diritto e a trovare le soluzioni alla domanda di giustizia dei cittadini.

non c'è bisogno! Si dice questi giovani prepareranno le minute delle sentenze e dei provvedimenti: non vorrei che invece si finisse per far scrivere le sentenze a questi giovani, perché in tal modo si violerebbe la Costituzione, o peggio ancora non vorrei invece che questi giovani venissero assunti per svolgere un lavoro intellettuale e finissero invece per svolgere un lavoro pratico all'interno delle cancellerie, dove c'è una cronica carenza di personale.

mancano 1.800 giudici. L'Italia non solo è uno dei Paesi in Europa che ha meno giudici per abitante, ma abbiamo anche un buco di organico di 1.800 magistrati, però ne abbiamo 250 distaccati nei Ministeri.

che volete mettere nell'ufficio del processo. Questo vorrebbe la logica, ma pretendere la logica in certi casi è davvero molto difficile. approfitto degli ultimi minuti che mi rimangono per parlare della magistratura onoraria.

Ovviamente ci siamo opposti a questo, perché è chiaro che i magistrati onorari meritano tutta l'attenzione che richiede la loro alta funzione giurisdizionale e soprattutto il loro senso di sacrificio e il loro senso delle istituzioni, perché hanno continuato a lavorare in condizioni assolutamente precarie, per garantire la giustizia anche in questi mesi così difficili di pandemia. Signori, dobbiamo però sottolineare con preoccupazione che il ministro Cartabia è gravemente inadempiente rispetto all'impegno, che aveva assunto, di formulare una proposta entro il 30 giugno. Siamo alla fine di luglio e non solo non c'è la proposta del ministro Cartabia, ma c'è una procedura di infrazione minacciata dalla Commissione europea

che in quella lettera è scritto che il Governo italiano sta calpestando il diritto dei lavoratori della giustizia onoraria, costretti a vivere e lavorare in un sistema di assoluto

Signor Presidente, mi dispiace dovermi ripetere per i colleghi di Fratelli d'Italia, però ci tengo davvero a ringraziare per la collaborazione che c'è stata

di poter andare in un altro ente nei Comuni con più di 100 dipendenti. Allo stesso tempo, garantiamo delle tempistiche adeguate affinché l'amministrazione comunale possa

Anche qui siamo riusciti ad approfondire veramente la questione e a trovare una soluzione. Oltretutto, questo si somma all'altro problema - che era già stato sollevato con un precedente provvedimento dei concorsi pubblici, che, secondo la nuova modalità istituita per il Covid, sono *on line* e hanno dei costi esorbitanti. La materia è stata comunque trattata, anche in questo caso, con il Ministero competente e sono felice di sapere che il ministro Brunetta,

Comuni, nel finanziamento di questi concorsi. Ringrazio anche il collega Manca, perché in Commissione ha presentato un emendamento, che abbiamo approvato, che dà la possibilità agli enti pubblici comunali di fare i concorsi in forma aggregata, diminuendo i costi. Quindi, vedete che ci sono anche colleghi che propongono cose giuste e occorre riconoscerle se vanno nell'interesse in questo caso delle amministrazioni comunali. Un altro punto su cui ci siamo battuti

e se un segretario non c'è, un Comune difficilmente potrà pensare al PNRR, se non riesce neanche a fare i Consigli e le Giunte comunali. *(Applausi)*. Vi è anche la possibilità di prorogare, da dodici a ventiquattro mesi, il tempo in servizio del vice segretario, visto che ci sono tantissimi Comuni in questo Paese, parlo in particolare della mia Lombardia, dove non c'è proprio un segretario. Quindi si prende tempo e si dà la possibilità di allungare questo periodo di sostituzione. Questo provvedimento, già nel suo testo base, è molto importante in quanto incarna l'auspicio di tanti giovani, che sono avvantaggiati come categoria per l'immissione nella pubblica amministrazione, di entrare a "svecchiare" i dipendenti pubblici, dando nuova linfa e freschezza anche al lavoro delle amministrazioni. Vi ricordo però che è giusto aiutare i giovani ad entrare nelle amministrazioni, ma in certe amministrazioni,

prima o poi risolvere: noi stiamo costruendo con questo decreto-legge e questo PNRR un bellissimo grattacielo di cinquanta piani, solidissimo, su delle fondamenta che scricchiolano; in questo caso parliamo degli enti territorialmente più vicini alla popolazione, che sono i Comuni. Stiamo mettendo risorse in termini economici e di personale

Io ho notato anche delle differenze di sensibilità tra i colleghi, che non rappresentano ovviamente la linea politica del loro partito, ma visioni personali, però sono stata molto amareggiata nel sentire alcuni colleghi che fuori onda o durante la Commissione hanno avuto espressioni infelici come "se un Comune piccolo non ha i soldi per aumentare lo stipendio ai propri dipendenti, può anche chiudere" o "i Comuni sono troppi". innanzitutto ci vuole rispetto quando si parla dei Comuni e dei nostri sindaci, categoria della quale io faccio orgogliosamente parte, soprattutto in questo periodo, dopo che, da oltre un anno, gestiscono la pandemia e stanno continuando farlo. In questi giorni, permettetemi di dare un grande abbraccio ai miei colleghi sindaci, alle loro popolazioni e a tutti i volontari che in tutta la penisola, all'acqua, al vento e al fuoco, si stanno adoperando per aiutare le loro popolazioni. *(Applausi)*. Ritengo, infatti, che nessuno qui abbia l'abitudine, nel tempo libero, di andare a spalare il fango, cosa che i sindaci normalmente fanno. Quindi, ci sono delle sensibilità

di ridare ai Comuni quello che è stato loro tolto negli ultimi dieci anni. I Comuni necessitano di soldi per le spese correnti, perché con i fondi del PNRR non si paga la corrente, non si paga il gas, non si paga l'acqua, non si pagano i dipendenti e non si pagano i servizi basilari ai cittadini. Ridiamo dignità ai Comuni, per favore - so di diventare noiosa, ma ve lo ripeterò fino allo sfinimento e più rispetto, perché il senso di comunità di questo Paese è quello dei Comuni. Penso, infatti, che a nessuno di voi farebbe piacere svegliarsi un giorno

Questo decreto viene mosso dall'esigenza di farsi trovare pronti alla sfida del *recovery plan*: un sacco di soldi che potremo avere se sapremo migliorare la nostra pubblica amministrazione e la nostra giustizia. Fin qui, ovviamente, siamo tutti d'accordo. Lo siamo meno, invece, su come farlo. Partiamo dalla questione Anac e dal fatto che uno Stato che deve spendere ingenti quantità di denaro deve anche essere in grado di controllare al meglio come viene impiegato questo denaro. Quindi, più soldi, più controlli. Da questo decreto, che mira a rafforzare la macchina pubblica, ci saremmo, pertanto, aspettati un rafforzamento dell'Autorità nazionale anticorruzione, con l'assunzione di nuovo personale, come infatti questo decreto prevede, giustamente, per tutte le altre pubbliche amministrazioni impegnate nell'attuazione del Piano nazionale. Purtroppo, questo non solo non è avvenuto, ma, al contrario, nel testo del decreto licenziato dal Consiglio dei ministri, l'Anac veniva di fatto indebolita. Nel tentativo, certamente giusto, di semplificare le procedure interne alle amministrazioni, il testo, tuttavia, rendeva incerta la funzione dell'Autorità anticorruzione nella lotta e nella prevenzione, appunto, della corruzione. Una problematica gigantesca, che, con non poca fatica, siamo riusciti a sanare. Vado a Nel testo originario il Dipartimento per la funzione pubblica (quindi, un pezzo del Governo) si sostituiva alle funzioni dell'Anac nei rapporti con le amministrazioni maggiori, quelle con più di 50 dipendenti. Come avveniva questo? diventando il soggetto preposto a redigere un piano tipo, che avrebbe contenuto anche le linee guida inviate all'amministrazione, proprio nell'ambito della trasparenza e dell'anticorruzione. Peccato che questo sia un compito di indirizzo proprio dell'Anac, attraverso il piano nazionale anticorruzione. Nonostante le avvisaglie e i moniti dell'attuale Presidente dell'autorità e, in maniera ancora più marcata, del suo predecessore, all'inizio pareva che nulla si muovesse: non nel Governo, ma, inizialmente, neanche all'interno delle Commissioni parlamentari, dove ben pochi, oltre a noi, sollevavano la questione. Eppure, quanto scritto in alcuni passaggi in alcuni passaggi dei testi di accompagnamento delle audizioni era chiarissimo. Raffaele Cantone dichiarava che la previsione dell'articolo 6, di un potere del Dipartimento funzione pubblica di adottare un piano tipo come strumento di supporto alle amministrazioni maggiori, finisce indiscutibilmente per interferire sui poteri che la legge attribuisce all'Anac. E ancora: il 30 giugno, il presidente Anac Giuseppe Busia dichiarava che una diversa allocazione di funzioni in materia di anticorruzione e trasparenza rischierebbe, innanzitutto, di non porsi in linea con la Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione. Con queste premesse l'ideale sarebbe stato cancellare la norma che creava questa interferenza del Governo nelle funzioni dell'Anac; un'interferenza generatrice di incertezza, proprio quell'incertezza che è tanto amata dai corrotti e dai corruttori. *(Applausi)*. Abbiamo presentato ovviamente l'emendamento soppressivo, ma non c'erano i numeri per approvarlo. Per fortuna, siamo riusciti comunque a rimettere le cose a posto facendo approvare un altro emendamento che chiarisce come le amministrazioni, nel redigere i propri piani anticorruzione, dovranno far riferimento alle linee guida dell'Anac e non alle linee guida di una parte del Governo che, a differenza dell'Anac, non è un'autorità indipendente. Mai avremmo permesso che in un periodo come questo, di impiego di enormi risorse economiche, si abbassasse la guardia nella lotta alla corruzione. poi la questione giustizia, dove si assumono a tempo determinato parecchie migliaia di persone per smaltire l'enorme mole di processi arretrati: scelta certamente positiva, decisa e pianificata dai Governi Conte, cui adesso si aggiunge il Piano previsto dal PNRR, ma in grado di sortire gli effetti sperati solo se ben impostata. Qui qualche preoccupazione c'è: basti ricordare il *flop* del recente concorso bandito dal Dipartimento della funzione pubblica per le assunzioni al Sud proprio per il *recovery* pochi partecipanti e assunzioni al palo, 821 su 2.800 posti messi a disposizione. Ci auguriamo che i decreti della Ministra della giustizia siano più efficaci di quello del Ministro per la pubblica amministrazione, ma anche qui qualche preoccupazione c'è se consideriamo i contenuti della cosiddetta riforma della giustizia che porta con sé enormi criticità. E non siamo solo noi a dirlo, ma lo dicono anche gli addetti al mestiere, coloro che operano negli uffici giudiziari; gente che vive le aule di giustizia con tutta la loro macchina amministrativa; persone che meritano di essere ascoltate per non incorrere nel tipico errore di presunzione di pensare che, per fare una riforma, basti conoscere la teoria appresa dai libri. Oltre alla teoria c'è la pratica, quella dei problemi che si vivono ogni giorno negli uffici giudiziari e che solo chi li frequenta e ci lavora può conoscere. Sono magistrati del calibro di Cafiero De Raho, il procuratore nazionale antimafia che addirittura ha parlato di un rischio per la sicurezza nazionale e la democrazia. Sono magistrati come Gratteri, Di Matteo, Scarpinato, Grasso, Caselli e tanti altri, magistrati e giuristi, con l'aggiunta - niente di meno - della bocciatura espressa dalla VI commissione del Consiglio superiore della magistratura nel parere che sarà discusso nel *plenum* e addirittura anche dall'Associazione nazionale magistrati. È in corso un'importante trattativa che vede impegnato tutto il MoVimento 5 Stelle con Giuseppe Conte: ce la stiamo mettendo tutta per migliorare il testo. Riteniamo che sia doveroso escludere dalla tagliola dei processi i reati più gravi, come quelli di mafia o di terrorismo; ma riteniamo anche che questo non possa bastare perché esistono molti altri reati, con pene ben al di sotto dell'ergastolo, che devono anch'essi essere esclusi dall'improcedibilità. Pensiamo - ad esempio - ai reati cosiddetti spia che portano spesso nelle braccia della mafia o dietro i quali essa si nasconde. Pensiamo alla corruzione o alle tante tipologie dei reati di violenza. L'Europa non ci chiede di cancellare i processi, ma di velocizzarli, di portarli a conclusione con una sentenza di condanna o di assoluzione. Il nostro deve essere uno Stato di diritto, non uno Stato di impunità; proprio quell'impunita che potrebbe giungere nonostante una sentenza di condanna in primo grado, secondo quanto previsto dalla proposta del Governo, per il solo fatto che sono scaduti i due anni per il processo di appello. Dire che, dopo due anni esatti dalla condanna in primo grado, il processo diventa improcedibile è come dire che il treno ad alta velocità Roma-Milano deve per forza impiegare tre ore esatte per completare il percorso e, se non lo dovesse fare, una volta scattate le tre ore, si ferma per sempre e fa scendere tutti i passeggeri, anche se si trova in campagna e nonostante i passeggeri abbiano pagato l'intero biglietto per un servizio che viene loro negato per una disposizione cervellotica. Quando avviene tutto questo? Qual è il contesto in cui tutto questo sta avvenendo? Esattamente nei giorni in cui sono state emesse condanne in appello per molti politici. Parlo dello scandalo denominato rimborsopoli Lombardia, che ha riguardato alcuni ex consiglieri regionali, tra cui l'attuale capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo; o ancora, delle condanne degli ex parlamentari di lungo corso di Forza Italia, Nicola Cosentino e Antonio D'Alì, anch'essi condannati in appello ma stavolta per reati ben più gravi. Tutti - ripeto tutti - questi politici oggi condannati in appello sarebbero rimasti impuniti se fosse già entrata in vigore la riforma Cartabia. È oggi il momento di parlare dei contenuti della proposta di modifica della nostra giustizia. Non ci sono ideologie o bandierine da sventolare; non deve esserci uno scontro tra politica e magistratura, come troppo spesso avviene in alcuni partiti. C'è e ci deve essere solo il bene esclusivo per il nostro Paese. È adesso che dobbiamo e possiamo evitare di risvegliarci un giorno quando sarà troppo tardi con centinaia di migliaia di processi cancellati. E sono convinto che siamo ancora in tempo per poterlo fare. *(Applausi)*.

Signor Presidente, approfitto di questa occasione non solo per ringraziare i relatori, senatori Valente e Caliendo, per il prezioso lavoro svolto, ma anche per

sono stati in alcuni momenti anche complessi e, quindi, anche gli Uffici hanno dovuto fare uno sforzo enorme, e credo di di rappresentare il sentimento di tutti nel dire che il loro supporto è stato assolutamente molto prezioso. Presidente, sono costretta a chiedere una sospensione dei lavori dell'Assemblea

l'orientamento è cambiato anche alla luce della complessità del provvedimento, delle votazioni e del lavoro che è stato svolto, per cui anche verificare nuovamente tutti i testi

che ora è alla Ragioneria generale dello Stato, ma ci vorranno delle ore per ricomporre le relazioni tecniche e bollinare il testo. Chiedo pertanto una sospensione dei lavori fino alle ore 19 di questa sera.

forse sarebbe il caso di fare una valutazione, alla conclusione del *question time*, del punto di arrivo del maxiemendamento.

prendo atto che la sua proposta è certamente migliorativa rispetto alla richiesta del Governo, ma mi consenta di esprimere il dissenso del Gruppo Fratelli d'Italia rispetto a tale richiesta, Grazie a tutti oltre al lavoro, abbiamo dovuto sopportare anche lunghe ed estenuanti interruzioni per le divisioni, le discussioni e, addirittura in certi casi, anche per le ripicche interne alla maggioranza, che il Sottosegretario conosce come

non solo che l'ennesima fiducia sia un *vulnus* inaccettabile per la dignità di quest'Aula, perché ormai è espropriata completamente di ogni potere e funzione di discutere nel merito. Diceva un collega poco fa che le leggi sono frutto della volontà generale, e non del Governo e dei voti di fiducia. Qui invece viene meno ogni confronto. È vero che in Commissione abbiamo avuto modo di svolgere alcune delle nostre considerazioni, ma in quest'Aula, come opposizione, avremmo il diritto di discutere sui provvedimenti, sugli emendamenti e anche di illustrare quei nostri pochi emendamenti che - come ci avete riconosciuto tutti - sono stati presentati nell'interesse di migliorare il provvedimento in discussione. Col voto di fiducia, tra l'altro, costringete l'opposizione a votare contro, quando invece avremmo avuto anche la possibilità, migliorando il testo, di arrivare a un voto non dico a favore, ma forse sì (o forse no, chi può saperlo). Da questo punto di vista, credo che in quest'Aula abbiamo diritto

fino alle ore 19 è veramente inaccettabile, ma anche la sua proposta, signor Presidente, è inaccettabile. Abbiamo diritto di conoscere subito quando sarà possibile iniziare la discussione e quando sarà possibile conoscere conoscere il testo definitivo e la relazione che deve accompagnare il maxiemendamento. La proposta che faccio è che alle ore 12,30 sì torni in Aula e il Governo ci dica esattamente i tempi che chiede al Senato Senato per poter proseguire nell'esame e con i nostri lavori. ieri la Commissione ha concluso i lavori alle ore 20. Il testo che raccoglie gli emendamenti approvati è stato trasmesso alle ore 4,15 di questa notte alla Ragioneria generale dello Stato relazioni tecniche. Non devo essere io l'avvocato della difesa d'ufficio, ma questi sono i numeri e i contenuti. La mia proposta è ovviamente anche di *moral suasion* rispetto alla Ragioneria, affinché lavori con la massima solerzia e ci consenta - speriamo speriamo nella giornata odierna - di poter approvare il provvedimento.

alle quali risponderanno il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della salute. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso. Avverto che, vista la coincidenza con il Consiglio dei ministri, modificheremo l'ordine

Signor Ministro, la ringrazio per il tempo che ci dedica oggi e per l'attenzione che vorrà riservare non solo alla situazione del trasporto e delle infrastrutture ferroviarie della Regione Piemonte, ma, più nello specifico, all'oggetto della mia interrogazione, che si focalizzerà su una questione relativa al mio territorio, ovvero Alessandria. La città di Alessandria rappresenta il Comune più esteso della Regione Piemonte e si trova al centro del triangolo industriale Torino-Milano-Genova, costituendo un importante nodo di interscambio. Storicamente la Provincia di Alessandria era dotata di un importante scalo merci ferroviario, il parco smistamento di Alessandria, un'area di oltre 500.000 metri quadri di proprietà di RFI e Mercitalia Rail, attualmente inutilizzata. Come sappiamo, nell'ambito della progettazione del Terzo valico, Alessandria è stata definita uno snodo importante e, nella legge di bilancio per il 2019, dall'allora ministro Toninelli

che si deve occupare della gestione del progetto. Ovviamente il polo alessandrino risulta essere un luogo scelto dai principali terminalisti come PSA, tra i *big* mondiali del settore logistico, per cui rientrerebbe a tutti gli effetti nel progetto più ampio della grande opera commissariata del Terzo valico. Ministro, fino ad oggi - e questa è la mia preoccupazione, su cui le chiedo qui conforto - al di là degli articoli di stampa, il parco smistamento non è rientrato né nelle opere da commissariare, né nei progetti del PNRR: è come se fosse scomparso dai radar. La mia domanda è quali siano i reali interessi, orientamenti e progetti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sull'area del parco smistamento di Alessandria; se sia possibile conoscere il cronoprogramma dei lavori, così come stabilito dall'accordo tra la UIRNet e RFI

l'intervento di progettazione del nuovo centro smistamento merci di Alessandria rientra tra le attività di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova, previste all'articolo 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e affidate al commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi, che ha provveduto a inserirlo nel programma straordinario di investimenti urgenti, approvato ai sensi dell'articolo 9-*bis* del medesimo decreto-legge. In data 19 luglio 2019 è stata sottoscritta, tra la struttura tecnica di missione del Ministero, l'autorità del sistema portuale del Mar Ligure occidentale e la società UIRNet, ora denominata DigITALog, una convenzione finalizzata a disciplinare le attività previste dal citato articolo 6. Detta convenzione riguarda anche la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria, per la cui realizzazione l'organismo di regia previsto dalla medesima convenzione ha stabilito: in considerazione dell'esistenza di infrastrutture ferroviarie, la sottoscrizione di un accordo tra UIRNet e RFI, per effettuare le attività di sopralluogo, analisi e progettazione dello scalo smistamento di Alessandria (l'accordo è stato sottoscritto in data 4 agosto 2020); la costituzione di uno *steering committee* di progetto, con la partecipazione di tutte le istituzioni coinvolte (detto organismo è stato costituito in data 21 maggio 2020); la definizione dei requisiti funzionali dell'area oggetto dell'intervento; l'effettuazione di una valutazione preliminare ambientale dell'area e l'eventuale sviluppo di un piano di modifica e, infine, la predisposizione di una progettazione di fattibilità tecnica ed economica, ivi compresa l'analisi costi-benefici. Al momento attuale, dei 2.000.000 di euro stanziati dalla legge di bilancio del 2019, per l'effettuazione delle attività di progettazione, risultano impegnati circa 165.000 euro, utilizzati dalla società DigITALog per la realizzazione dello studio trasportistico propedeutico all'elaborazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica da parte di RFI, in attuazione del citato accordo. DigITALog riferisce che lo studio trasportistico si concluderà nei primi giorni del prossimo mese di settembre. Quanto al ripristino degli storici collegamenti ferroviari per l'utenza pendolare, Ferrovie dello Stato ha comunicato che è in corso la necessaria attività di analisi della domanda di trasporto, la cui conclusione è prevista per la fine del mese di agosto. Al termine di questi due passaggi saremo quindi in grado di avviare i passaggi successivi.

alle due grandi opere: Terzo valico e TAV - si parla sempre di arricchimento dei territori, di nuovi posti di lavoro e si parla di Alessandria come naturale retro-porto di Genova e quindi di supportare il decongestionamento delle aree urbane tramite lo spostamento del traffico da gomma a rotaia. Questo è importante, soprattutto

di nuovo centrale e quindi non più marginale, per tutto il Piemonte e l'Italia intera. Chiedo celerità perché, quando si parla di soldi dei cittadini, fossero anche 1.000 euro,

*(Aut (SVP-PATT, UV))*. Egregio Ministro, la certificazione verde Covid-19 rende più semplice viaggiare da e verso tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen. In Italia la certificazione verde serve per partecipare alle feste, per cerimonie civili e religiose, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, nonché per spostarsi in entrata e in uscita dai territori classificati in zona rossa o arancione. L'articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, prevede che, a far data dal prossimo 6 agosto, la certificazione verde servirà per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici. Stante le informazioni ricevute dall'azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, sembra che circa 70.000 persone che hanno effettuato la vaccinazione anti-Covid, pur avendo ricevuto dalla Provincia il certificato vaccinale Corona *pass*, lamentino di non aver ricevuto a tutt'oggi il codice *authcode* per accedere al proprio *green pass*. Le richieste del codice *authcode* da parte degli interessati sono state sollecitate, ma senza successo, secondo le indicazioni disponibili sul sito del Ministero della salute, ossia contattando il numero 1500 o con *e-mail* indirizzata all'indirizzo di posta elettronica. La Provincia autonoma di Bolzano trasmette con regolarità alla piattaforma nazionale i dati delle persone vaccinate contro il Covid-19, di quelle guarite e di quelle che hanno ottenuto un risultato negativo al *test* molecolare antigenico. l'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano ha già richiesto, con urgenza, in data 20 luglio, al Ministero una serie di informazioni tecniche e proposto diverse soluzioni per risolvere il problema lamentato, si chiede di sapere, vista la crescente preoccupazione delle persone che non hanno ancora ottenuto il *green pass* e che dal 12 agosto 2021 non potranno più neanche utilizzare l'attestato di vaccinazione emesso dal servizio sanitario locale per accedere ai servizi menzionati o per viaggiare, quali siano le motivazioni che ostacolano il suo rilascio, i tempi necessari e le modalità per risolvere il problema.

il tema del *green pass* che il Governo ritiene essere un pezzo essenziale della strategia di gestione di questa fase epidemica, che è diversa proprio perché caratterizzata da un'alta percentuale di persone vaccinate nel nostro Paese. Riteniamo che il *green pass* sia uno strumento molto importante che può aiutarci a rendere più sicuri i luoghi in cui esso è applicato e che ci aiuterà sicuramente a limitare le restrizioni.

Paese. Vengo velocemente ai numeri della Provincia di Bolzano, per come mi vengono riportati dai nostri uffici. Nella Provincia di Bolzano sono stati emessi 499.874 *green pass*, di cui 51.242 per tampone, 48.995 per guarigione e 399.637 per vaccinazione. La Provincia di Bolzano ha trasferito alle autorità nazionali 265.870 *e-mail* che sono state utilizzate per l'invio dell'*authcode* e 96.910 numeri di telefono a cui è stato mandato l'SMS. Restano circa 36.850 persone

mi piace informare l'Assemblea del Senato che a breve sarà possibile, anche attraverso il sito, avere un meccanismo di generazione automatica dell'*authcode* che renderà ancora più semplice la procedura. Confermo, in conclusione, che è intenzione del Governo continuare a investire in questo strumento, che riteniamo davvero importante per la gestione di questa stagione epidemica.

lo Stato deve fare la sua parte, sia in merito all'organizzazione della vaccinazione, sia in merito al rilascio tempestivo della certificazione verde. In merito a quest'ultimo aspetto, sono 70.000 le persone che mi vengono segnalate dell'Azienda sanitaria locale (lei parla di 36.000 persone) che aspettano, ormai da settimane e alcuni da mesi, questo certificato verde nella sola Provincia autonoma di Bolzano: sono davvero troppe. Quindi auspico che, soprattutto i problemi tecnici che mi vengono segnalati possano essere risolti in tempi brevi e che ciò comporti un miglioramento della situazione. In attesa

dei certificati verdi e sui fenomeni di contraffazione, per il Ministro - intende preservare noi stessi e gli altri dal contagio, proteggere le attività economiche, evitando altre chiusure, e difendere la campagna vaccinale che sta andando molto bene, con un'adesione massiccia dei giovani. Siamo contenti per la responsabilità dei cittadini. Proprio per questo le chiedo, Ministro, se e come intende organizzare un monitoraggio più preciso di alcune criticità che i nostri cittadini ancora incontrano: non sempre si riesce a ricevere il codice per la generazione del *green pass* in tempi tempestivi; occorre un'attenzione in più a chi è guarito dal Covid Covid e non è riuscito ad ottenere il *green pass* (mi pare che su tutto il territorio nazionale sia in gran parte risolto questo problema, ma non è sempre così).

del 23 luglio 2021. Sappiamo che Il Ministero ha fatto tanto anche per evitare la contraffazione dei *green pass*. C'è un'*app* come intenda comunicare queste iniziative alla cittadinanza, che spesso non ne è a conoscenza. Un ultimo argomento che ci sta particolarmente a cuore è l'accesso dei parenti alle strutture ospedaliere e come si intenda si intenda concretizzare il decreto del 23 luglio ha ampliato la possibilità di ingresso dei parenti - e di questo siamo contenti - ma dobbiamo giungere alla possibilità per i parenti dei pazienti ricoverati di arrivare anche ai reparti, naturalmente in estrema sicurezza, perché credo che la presenza del familiare del paziente sia essenziale per la cura delle malattie.

di provare a limitare il più possibile le restrizioni in una fase diversa dell'epidemia, perché l'epidemia è ancora in corso, ma avendo numeri di vaccinazione ormai molto significativi, con lo strumento del *green pass* possiamo provare a costruire una strategia diversa. Come già dicevo, questi numeri sono significativi di

al giorno. La nostra macchina è al lavoro anche per intervenire in modo più puntuale su specifiche fattispecie ove dovessero esserci delle difficoltà. Credo sia particolarmente significativa

la presenza e l'ausilio delle farmacie e dei medici di medicina generale, le numerose modalità messe in campo hanno consentito un risultato che, sinceramente, è davvero molto importante. Sui punti specifici che si ponevano, anche rispetto all'AIRE, c'è un lavoro in corso. Mi auguro che, all'inizio della prossima settimana, questo lavoro potrà portare a una soluzione definitiva. Sulla vicenda delle RSA, dei presidi ospedalieri e dei reparti ospedalieri, l'articolo 4 del decreto-legge n. 105, approvato in Consiglio dei ministri giovedì, giovedì, estende la disposizione che, per la verità, io avevo assunto, con mia ordinanza, l'8 maggio per le RSA e che poi il Parlamento, in sede di conversione di un precedente decreto,

ma anche per l'accesso ai reparti ospedalieri. Questo gruppo di lavoro dell'Agenas, costituito con le Regioni, ha esattamente la finalità di monitorare che questo diritto venga pienamente esercitato da parte di tutti.

che dobbiamo aver cura degli altri e dei più fragili. Quindi, dobbiamo scrivere delle norme. Il Parlamento farà la sua parte adesso che arriva il decreto-legge che lei citava. Dobbiamo scrivere norme più stringenti e direttive chiare perché queste vengano attuate e aiutare le strutture sanitarie, le Regioni e le ASL a permettere ai familiari di essere vicino ai parenti in un momento di fragilità. Dobbiamo uscire da questa epidemia con una grande solidarietà

Ministro, noi abbiamo delle perplessità che le illustriamo. La prima riguarda l'eventualità che il Ministero intenda procedere alla vaccinazione, che viene definita di massa, e, quindi, intenda raccomandare alle Regioni di spingere sulla vaccinazione ai dodicenni e ai tredicenni, nonostante esistano nella comunità scientifica ampie fasce di dubbio rispetto alla possibilità alla possibilità di quantificare il famoso costo beneficio di questa vaccinazione, cioè i possibili problemi derivanti da una vaccinazione di una persona che ha davanti un'aspettativa di vita di circa settant'anni.

gratuiti per docenti, personale ATA e studenti, implementare le sedi scolastiche per evitare le cosiddette classi pollaio, regolare il trasporto pubblico locale per garantire il trasporto in sicurezza sicurezza e trovare soluzioni di conciliazione degli orari di lavoro dei genitori per incentivare l'utilizzo dell'auto privata per portare i ragazzi a scuola. Di tutto questo non c'è traccia, Ministro, aspettiamo di conoscere la sua risposta. Sono domande che si

ringrazio gli interroganti per l'occasione di chiarire che per il Governo la campagna di vaccinazione è davvero lo strumento fondamentale per chiudere questa stagione così difficile. I numeri italiani sono davvero molto incoraggianti e credo siano patrimonio di tutto il Paese, senza alcuna distinzione. A stamattina abbiamo somministrato

Anche nella fascia di età tra i dodici e i diciannove anni i numeri sono incoraggianti. Infatti, nonostante questa vaccinazione sia iniziata molto più tardi nel tempo, il 30 per cento delle persone vaccinabili in quella fascia d'età ha ricevuto una prima dose e il 15 per cento anche la seconda. Come

in questi mesi così difficili, ritiene che scelte di questa natura debbono avere fondamento di evidenza scientifica. Noi abbiamo fiducia nelle nostre istituzioni internazionali, l'EMA, da una parte, e l'AIFA, dall'altra. L'AIFA, tra l'altro,

La nostra comunità scientifica nazionale, che su questa materia si è lungamente confrontata, ha espresso un'opinione favorevole su tale vaccinazione; lo ha fatto il nostro Comitato tecnico-scientifico, di cui fa parte il presidente del consiglio superiore di sanità, che ha più volte fatto dichiarazioni in tal senso, il presidente dell'Istituto superiore di sanità e il presidente dell'AIFA stessa. Anche la Società italiana di pediatria, con un'espressione di natura formale, ha raccomandato la vaccinazione. Le ragioni fondamentali sono due: la prima è che la vaccinazione protegge chi riceve il vaccino. Anche in questa fascia purtroppo ci sono casi di persone che contraggono il virus con una conseguente situazione di gravità. Abbiamo visto, purtroppo, in un fatto di cronaca molto recente, delle ultime ore, nella città di Palermo, in Sicilia, come una bambina di undici anni abbia addirittura perso la vita. la vita. Inoltre, chi si vaccina non protegge solo se stesso ma aiuta la protezione di tutti gli altri e non vi è alcun dubbio che anche una vaccinazione all'interno di quella fascia generazionale potrà favorire la riduzione della circolazione del virus. Questo tema è ancora più vero se pensiamo al secondo ambito dell'interrogazione che mi viene rivolta, cioè quello delle scuole. Siamo al lavoro per costruire modalità che ci consentano una ripresa e una ripartenza in presenza e in sicurezza. Questo è l'obiettivo del Governo. Il nostro Ministro dell'istruzione ha aperto un confronto con le parti sociali, con i sindacati, con tutte le variegate rappresentanze del mondo della scuola. C'è una discussione aperta anche con le Regioni e il Governo sicuramente non farà mancare un'iniziativa molto forte anche su questo tema per raggiungere un obiettivo che consideriamo assolutamente strategico. Ministro, siamo soddisfatti dei numeri che ci illustra sulla campagna vaccinale, perché Fratelli d'Italia è un partito *pro* vax. Detto questo, ci facciamo delle domande alle quali ci piacerebbe venisse data una risposta seria. siete sicuri che non esistono problemi a vaccinare un dodicenne, togliete dal consenso informato la frase che dice che non siamo in grado di prevedere quali sono gli effetti a lunga scadenza.

Grazie a tutti oggi o domani, ma ieri, perché mancano quaranta giorni all'apertura della scuola e per adottare provvedimenti seri e reali non abbiamo il tempo materiale di farlo. Dovevate licenziare oggi il piano scuola; avete ulteriormente rimandato. La sensazione evidente,

È evidente la volontà di scaricare sui cittadini, quindi con ulteriori restrizioni delle libertà di impresa e individuali, i ritardi e le inadempienze dello Stato e del Governo. Fratelli d'Italia è un partito *pro* vax,

che questi dati facciano riflettere tutti. Si esca dalle narrazioni inutili e dannose, così magari riusciamo tutti a stringerci attorno alla sintesi intelligente e responsabile che ha fatto il Presidente della Repubblica: chi limita le nostre libertà è il virus, non gli strumenti per sconfiggerlo. Colleghe e colleghi, l'elemento della chiarezza e della nettezza, senza ambiguità, sulla questione dei vaccini e della gestione della campagna vaccinale è una responsabilità di tutti noi, non solo del Governo o del generale Figliuolo. Gli italiani hanno bisogno di chiarezza e purtroppo a volte non c'è. Rivolgo una domanda precisa al Ministro. Sulla scuola e sui trasporti bisogna assolutamente accelerare. Sinceramente non mi convince quest'ultimo rinvio; dobbiamo articolare gli orari e fare una scelta sugli insegnanti e sul *green pass* e dobbiamo risolvere il problema dei trasporti. Non possiamo scoprire fra un mese che questi problemi non sono risolti. La DAD non può essere la risposta: la scelta di tutti noi è in presenza e questo richiede interventi straordinari e, da parte di tutti noi, la cessazione di messaggi ambigui. La vaccinazione è decisiva.

I numeri riportati dalla fondazione Gimbe, ma anche dal nostro *report* settimanale a cura dell'Istituto superiore di sanità, sono molto chiari e rispecchiano una tendenza che evidentemente non è solo italiana: nel quadro europeo nel quadro europeo c'è un aumento consistente del numero di persone contagiate quotidianamente. La causa è presto detta: una nuova variante, la variante Delta, ha una capacità di contagiare molto più significativa rispetto alla variante Alfa, che era prima dominante. L'attesa dei nostri tecnici e dei nostri scienziati è che la variante Delta, da qui al mese di agosto, diventerà dominante in tutti i Paesi europei, compreso naturalmente il nostro. Dentro questo quadro, l'arma in più che abbiamo è sicuramente quella delle vaccinazioni. Dicevo che siamo arrivati a 67 milioni di dosi somministrate, che è un dato straordinariamente positivo. Siamo al 66 per cento di prime dosi sulla popolazione vaccinabili e al 58 per cento di seconde dosi sulla popolazione vaccinabile. Dobbiamo continuare ed insistere su questo terreno. È chiaro che la campagna di vaccinazione è la vera arma di libertà che abbiamo e che può consentirci di evitare quelle chiusure che abbiamo conosciuto in altri momenti e in altri tempi. Non vi è alcun dubbio, senatore Errani, che la questione scuola è per il Governo una questione assolutamente prioritaria. Sono fiducioso che la prossima settimana sarà quella giusta per un intervento più organico che ci consenta di programmare una ripartenza che tutto il Governo vuole che sia in presenza e in sicurezza (questi due aspetti devono tenersi insieme). Vogliamo lavorare perché i nostri ragazzi e i nostri figli possano tornare a scuola in presenza, superando quindi una lunga stagione di didattica a distanza, ma anche in sicurezza, e utilizzeremo tutti gli strumenti possibili per realizzare questo obiettivo. Voglio ricordare che l'85 per cento del personale scolastico scolastico ha già avuto una prima dose (una cifra assolutamente considerevole), e il Governo lavora perché questa percentuale possa ancora crescere in maniera molto significativa. Ringrazio per l'interrogazione e penso che su questi temi tutto il Parlamento dovrebbe condividere, dal mio punto di vista, lo spirito espresso ieri nelle parole del Presidente della Repubblica, che condivido profondamente.

non vogliamo più arrivare ai *lockdown*. Per fare questo occorrono tre condizioni: campagna vaccinale senza ambiguità; tracciamento, utilizzando anche le piattaforme che ci garantiscono il tracciamento, poiché oggi abbiamo numeri che ci consentono tale tracciamento per limitare e isolare i casi; sequenziamento sulle variazioni del virus. Questo è un impegno su cui dobbiamo assolutamente riuscire a fare un salto di qualità anche in relazione ai problemi che Immuni

Premesso che: negli ultimi mesi si sono susseguiti numerosi tragici fatti di cronaca: a Trevignano romano (Roma) dove un giovane con problemi di tossicodipendenza ha ucciso la madre e la vicina, e successivamente ha investito

con all'interno il coltello da cucina, spiegando che si era mosso con l'intenzione di uccidere qualcuno; a Bolzano, dove un giovane ha ucciso entrambi i genitori, riportando di soffrire di un disturbo del sonno; o, ancora, il caso di Ardea (Roma), dove un uomo, già noto per i suoi problemi psichiatrici, ha ucciso due bambini e un anziano preso da uno scatto d'ira e, da e, da ultimo, ma non certo ultimo, il caso del ragazzo di 16 anni di Monteveglio (Bologna) che ha assassinato l'amica coetanea dichiarando di aver sentito dei demoni che lo hanno spinto alla violenza; questi fatti hanno fatto riemergere il problema, mai sopito, in ordine all'assenza di strutture adeguate preposte alla cura e al supporto di quanti soffrono di problemi psichici e delle loro famiglie; caposaldo della legislazione nazionale in tema di salute mentale è la legge 13 maggio 1978, n. 180, nota anche come "legge Basaglia", dal nome del suo promotore, che ha disposto la chiusura degli ospedali psichiatrici, predisponendo un sistema di assistenza psichiatrica facendo così emergere l'incapacità del comparto pubblico di salute mentale a soddisfare la domanda di coloro che sono affetti da disturbi e che non hanno le possibilità economiche di rivolgersi a strutture private e in generale la mancanza di un'adeguata assistenza alle famiglie; sono diverse le associazioni dei familiari e delle persone che vivono l'esperienza del disturbo mentale che denunciano l'inadeguatezza della rete dei servizi di salute mentale, richiedendo una maggiore attenzione e risposte concrete, in ordine alle conseguenze legate alla convivenza con persone affette da disturbi, in special modo in riferimento all'incolumità personale in caso di un disturbo di personalità grave del malato,

e protezione del malato, di sostegno alle famiglie, nonché di prevenzione dei reati. ringrazio molto gli interroganti per aver voluto porre l'attenzione su un tema che considero assolutamente centrale e strategico per il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale, qual è quello della salute mentale. Mi sia permesso in premessa di esprimere gratitudine per le donne e gli uomini del Servizio sanitario nazionale che lavorano nei dipartimenti di salute mentale, perché svolgono ogni giorno un lavoro straordinario, spesso in condizioni non facili, così come desidero esprimere gratitudine alle reti di volontariato e del terzo settore che lavorano quotidianamente a supporto dei dipartimenti di prevenzione. Voglio ricordare all'Assemblea che proprio il 25 e il 26 giugno di quest'anno ho promosso la Conferenza nazionale sulla salute mentale, che nel nostro Paese non si teneva da vent'anni ed è stata una grandissima occasione per rilanciare una stagione di nuovi investimenti. Questo appuntamento, aperto da due messaggi autorevolissimi come quelli del Presidente della Repubblica e del Santo Padre, Papa Francesco, e che ha visto la partecipazione anche dei Ministri del lavoro e della giustizia, che hanno competenze molto forti proprio per le ragioni a cui si faceva riferimento nell'interrogazione, è stato a mio parere un appuntamento importante che ci consente ora di pianificare una nuova fase di investimenti. Voglio, tra l'altro, ricordare, proprio a riprova di come consideriamo questo tema fondamentale, che anche durante il G20, di cui l'Italia come è noto quest'anno ha la Presidenza, ci sarà un *side* *event* esattamente sulla salute mentale. L'Italia ha una grande tradizione in questo campo, in termini di attenzione alle tematiche della salute mentale: dalla legge Basaglia in poi, che è stata una norma di grandissima civiltà che ha qualificato il nostro Paese anche a livello internazionale, sono stati molti i provvedimenti costruiti che ci hanno consentito di elaborare anche una buona pratica guardata con attenzione a livello internazionale. Nell'interrogazione si pone un tema che condivido e cioè quello della disparità della qualità dei servizi di salute mentale offerti in ambito regionale diverse aree del nostro territorio, un grande tema su cui dobbiamo lavorare e dobbiamo investire. Questo è l'impegno del Governo. Lo faremo con nostre risorse con nostre risorse nazionali, penso ad esempio, per quanto mi riguarda, alle risorse dell'edilizia sanitaria *ex* articolo 20 della legge del 1988, ma sto lavorando anche perché risorse comunitarie importanti possano essere utilizzate esattamente per questo tentativo. In conclusione, voglio garantire, anche alla luce delle cose che ho velocemente enunciato, che c'è la massima attenzione del Governo e che considero personalmente la questione del rafforzamento dei nostri dipartimenti di salute mentale una questione prioritaria su cui mettere il massimo impegno come Governo.

In quasi tutti i Paesi del mondo sono rimaste attive strutture ospedaliere per la cura dei pazienti affetti da disturbi psicotici, che non hanno consapevolezza della malattia e che presentano scarsa In Italia invece, nonostante quanto previsto dall'articolo 32 della Carta costituzionale, tale possibilità di cura è negata dalla legge anche per i pazienti che volontariamente richiedono di essere curati e ricoverati. Perché? Attenzione al paradosso: sebbene il malato di mente oggi sia ritenuto non più pericoloso per sé stesso e per gli altri, ma solo bisognoso di assistenza, paradossalmente è ancora possibile disporre di misure restrittive della libertà personale mediante il ricovero coatto, il TSO è un provvedimento rigido e complesso. Nel corso degli ultimi decenni l'offerta psichiatrica si è trasformata in banale assistenzialismo, alimentando tra l'altro la paura per la riapertura dei vecchi manicomi. Ministro Speranza, mi perdoni, il vecchio modello manicomiale con elettroshock e bagni gelidi sta come i salassi e le sanguisughe alla moderna cardiochirurgia. *(Applausi)*. alle richieste della Lega nello specifico non è stata presa alcuna posizione sulla necessità della modifica della legge n. 180 per offrire dignitose e doverose cure mediche non assistenziali ai pazienti psichiatrici e alleggerire le famiglie, da cui si leva un urlo silente che - le assicuro

ha destituito di fatto il Capo del Governo e ha inviato l'esercito presso le sedi del Parlamento e del Governo, invocando l'articolo 80 della Costituzione. Al netto delle disquisizioni che potremmo fare sul perimetro di un articolo della Costituzione di uno Stato estero, preme a noi esprimere delle preoccupazioni e chiedere quali sono le iniziative che intendano mettere in campo il Ministero degli affari esteri e il Governo nelle sedi europee e nelle sedi internazionali per ciò che succede a pochi chilometri dalle nostre coste. Ricordo, infatti, che Pantelleria è a pochi chilometri da Tunisi e a pochi chilometri dalle coste siciliane. tunisina preoccupa da un po' di tempo dal punto di vista economico, con un calo del reddito *pro capite* negli ultimi dieci anni del 34 per cento, evidentemente acuito dalla crisi del Covid. Ad essere coinvolto è, in particolare, il settore turistico, che costituisce un'ossatura importante del sistema economico tunisino non c'è bisogno di dire come la crisi economica in un Paese così vicino si riverberi nei confronti dell'Italia, cui la Tunisia è legata da rapporti commerciali e culturali di forte integrazione, soprattutto tra le comunità delle Regioni del Sud.

dunque preoccupati per una situazione che ci deve vedere protagonisti per la stabilità del Mediterraneo centrale, di un Paese così importante per il nostro territorio. doverci trovare ad affrontare nuove situazioni post-primavere arabe, motivi per cui i tentativi di costruire percorsi democratici nei Paesi del Nord Africa incontrino uno stop che rischia di riverberarsi poi anche sulla politica estera del nostro Paese e dei Paesi del Mediterraneo. La situazione in Tunisia è fonte di forte preoccupazione. Seguiamo con la massima attenzione gli effetti delle decisioni assunte dal presidente della Repubblica Saïed nella notte fra il 25 e il 26 luglio. Nelle ore successive all'annuncio del Presidente abbiamo subito dato un forte impulso per avviare un coordinamento con i principali *partner* europei. Nella convinzione che l'Unione europea possa

poi concretizzatasi nella pubblicazione del comunicato a nome di tutti e 27 gli Stati membri sulla situazione in Tunisia. Ieri ho discusso delle vicende tunisine anche con il ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian. Da tutti questi colloqui, così come dalle interlocuzioni a livello di funzionari, emerge unanime la necessità di ribadire alle istituzioni tunisine un forte appello alla responsabilità e al rispetto della democrazia e dello stato di diritto. La Costituzione tunisina deve essere pienamente rispettata. Occorre consentire al Parlamento legittimamente eletto di svolgere le proprie funzioni. Sono questi i messaggi che ho trasmesso sempre ieri al ministro degli affari esteri tunisino, Othman Jerandi, nel colloquio telefonico che abbiamo avuto. Al collega di Tunisi ho anche rinnovato l'appello alla moderazione, affinché venga presa ogni iniziativa per evitare scontri e violenze. Il Ministro degli affari esteri mi ha assicurato che la Costituzione verrà rispettata, ha aggiunto che il Presidente sta svolgendo consultazioni per nominare a breve un nuovo Primo ministro e che sarà poi tempestivamente affrontata la questione della ripresa del Parlamento Gli sviluppi degli ultimi giorni intervengono in un momento molto complicato per la Tunisia, già attanagliata da una gravissima crisi economica, a cui si è aggiunta l'emergenza pandemica. Le difficoltà incontrate dal Governo tunisino all'avvio dei negoziati con il Fondo monetario internazionale, per un nuovo programma di aiuti finanziari, si sono infatti intrecciate con l'aggravarsi del quadro epidemiologico. In conclusione, signor Presidente, l'Italia rimane determinata a garantire il proprio sostegno alla Tunisia, nel complesso del dialogo con il Fondo monetario internazionale, passaggio fondamentale per permettere l'attuazione di riforme economiche necessarie. Intendiamo mantenere lo stesso impegno nella collaborazione sul fronte del contrasto all'epidemia. Dopo i cinque *container* di materiale sanitario e le donazioni per l'acquisto di generatori di ossigeno per gli ospedali tunisini, nei prossimi giorni l'Italia donerà alla Tunisia una scorta di vaccini. Non faremo mancare il nostro sostegno a un popolo da sempre amico e continueremo a lavorare con l'Unione europea per favorire la stabilità e la democrazia in Tunisia, Paese che sentiamo non solo vicino, ma partecipe di un destino comune.

nell'azione mirata a verificare il rispetto delle condizioni garantite dalla Costituzione, perché possa riprendere l'attività parlamentare e garantire il percorso democratico che è avvenuto dopo la rivoluzione dei gelsomini, che ha portato a un'esperienza senza eguali nel Nord Africa. Colgo l'occasione per rimarcare la preoccupazione invece rispetto ad altri teatri, dove magari l'esigenza di *Realpolitik* e di garantire la stabilità è andata verso forme di Governo che non danno garanzie del rispetto dei più elementari diritti umani. Quindi la nostra preoccupazione è che si concilino la stabilità e la sicurezza di un Paese, per noi fondamentale per la vicinanza e i rapporti che abbiamo, con la possibilità di accompagnare le migliori esperienze democratiche, affinché non si interrompano e non contribuiscano a creare instabilità, in un'area per noi strategica, come quella del Mediterraneo.

fatti gravissimi, con una popolazione ridotta allo stremo: non ci sono i generi di prima necessità, sono alla fame e non basta nemmeno più la *libreta*, la tessera che

con un mare pescoso, che potrebbe garantire aiuto anche ad altri o comunque a tutta l'isola. Eppure, proprio quel regime comunista è arrivato ad affamare il proprio popolo, che è sceso in è sceso in piazza, come sapete tutti, qualche giorno fa, a rischio anche della propria vita. Ci sono stati morti e feriti e alcune persone sono state addirittura prelevate e deportate nei campi di concentramento, che pure esistono a Cuba, e anche nei campi di lavoro. Ci sono famiglie distrutte e *desaparecido*. È una situazione difficile: sono state usate violenze e perquisizioni arbitrarie. un popolo in ginocchio e, là dove c'è un popolo in ginocchio, Forza Italia, ma penso di poter dire tutto il centrodestra e mi auguro tutta l'Assemblea, vogliono essere presenti, per dare solidarietà e soprattutto risposte risposte importanti. Ecco perché ci siamo permessi di rivolgerle alcune domande importanti, anzitutto per sapere qual è la sua posizione, signor Ministro, che è ovviamente quella del Governo, e se si intenda manifestare pubblicamente solidarietà al popolo cubano e, con egual forza e in egual misura, nei confronti del Governo cubano che sta affamando quel popolo. Soprattutto, le chiediamo di convocare l'ambasciatore cubano a Roma,

essere attuato un piano di interventi a Cuba, accompagnato da alcune garanzie, come la libertà di manifestare. Liberazione dei detenuti politici, libertà di manifestazione e ritorno della democrazia in quelle terre: questo è quello che le chiediamo e ci aspettiamo una risposta adeguata

senatori, ringrazio il senatore interrogante. Le manifestazioni svoltesi sia Cuba l'11 luglio scorso hanno visto un'ampia partecipazione della popolazione. Si è trattato di una delle dimostrazioni più significative dal 1994 Da decenni il Governo mantiene un approccio restrittivo e repressivo riguardo ai diritti civili e politici e alle libertà fondamentali dei propri cittadini. A scatenare la protesta sono state soprattutto la grave crisi economica ed energetica, la carenza di generi alimentari di prima necessità e l'impennata dei contagi da Covid, che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario cubano, nonostante l'intensificarsi della campagna vaccinale. Le manifestazioni hanno fatto registrare una vittima, decine di feriti e numerosi arresti di persone ritenute dalle autorità cubane agitatori per conto di attori esterni. L'Avana accusa infatti gli Stati Uniti, che mantengono un duro embargo nei confronti del Paese, di fomentare le proteste per violare la sovranità dell'isola e rovesciare il regime. Il Direttore generale per la mondializzazione e le questioni globali del Ministero degli affari esteri ha incontrato l'ambasciatore cubano a Roma il 13 luglio. In questa occasione abbiamo espresso tutta la nostra preoccupazione per la gestione dell'ordine pubblico e delle persone fermate. Abbiamo inoltre chiesto adeguata protezione per i cittadini italiani eventualmente coinvolti nelle dimostrazioni e per la nostra sede diplomatica, qualora le circostanze lo rendessero necessario. È essenziale che venga pienamente rispettato lo Stato di diritto e per questo abbiamo sostenuto l'appello dell'alto rappresentante dell'Unione europea Borrell affinché sia consentito al popolo cubano di manifestare liberamente. Le persone fermate devono essere adeguatamente giudicate, se ritenute responsabili di reati durante le dimostrazioni, oppure immediatamente rilasciate, in caso di mancanza di prove. Lavoriamo per favorire nel Paese il riconoscimento e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a partire dalla libera manifestazione del pensiero. Perseguiamo quest'obiettivo sul piano bilaterale nell'ambito del meccanismo di dialogo politico istituito nel 2011 e riunitosi più volte e nel più ampio contesto europeo, in collaborazione con il Servizio europeo per l'azione esterna. Il dialogo sui diritti umani tra Unione europea e Cuba è uno strumento ormai ben rodato rappresenta la cornice migliore nell'ambito della quale proseguire il confronto con le autorità cubane. Alla nostra ferma posizione politica associamo un costante impegno a favore della popolazione cubana. Da dieci anni, Cuba è un Paese prioritario per la nostra cooperazione allo sviluppo. Fin dall'inizio della pandemia, abbiamo riorientato alcune delle attività per far fronte all'emergenza sanitaria alle sue ripercussioni socio-economiche. Sul canale umanitario sosteniamo le attività del Programma alimentare mondiale, in particolare per la fornitura di generi alimentari a oltre 2.000 pazienti ricoverati per Covid in sette strutture ospedaliere del Paese. L'Italia è al fianco del popolo cubano nella sua ricerca di un futuro migliore in termini di libertà e benessere. Signor Ministro, dobbiamo far sentire alta e forte la voce dell'Italia e soprattutto della comunità internazionale e dobbiamo aiutare il popolo cubano. Il presupposto,

di quale livello di violenza sto parlando. Forza Italia si è battuta, signor Ministro, in questi ultimi anni per battaglie di libertà: a Cuba, naturalmente, come stiamo facendo in questo momento, ma anche in Nicaragua e in Venezuela, così come ad Hong Kong. Là dove c'è il comunismo, purtroppo i regimi comunisti stanno dimostrando di essere una tragica infezione, anche della politica.

ma abbiamo sentito intorno a noi un silenzio anecoico, molto spesso da parte della stampa. Infatti, è molto facile fare i comunisti in un Paese libero, ma è più difficile essere liberi in un Paese comunista. Questa è la ragione per la quale noi di Forza Italia, ma credo di poter dire gran parte di quest'Assemblea, siamo dalla parte della libertà e continueremo ad esserlo.

iniziò proprio in quest'Aula del Senato, il 23 gennaio 2019, una campagna calunniosa e diffamatoria, amplificata anche da parte di colleghi che ben conoscevano la mia storia trentennale a tutela dei diritti e della legalità contro ogni discriminazione di classe, razza e religione, meglio conosciuta come odio razziale. Una gogna mediatica che ha coinvolto anche la mia famiglia e che ho subìto in silenzio per quasi trenta per un *tweet* sui Savi di Sion, prontamente rimosso il giorno dopo con relative scuse, ma andata avanti per mesi su *talk show*, TV, radio e *mass media*, dopo la querela del Presidente della comunità ebraica, che aveva denunciato quel *post* sui *social* *media* del 20 gennaio 2019. Patrocinato gratuitamente dal professor Astolfo Di Amato, che ringrazio, perché conosceva la mia storia, la procura di Roma il 5 febbraio 2020 ha rilevato che le mie affermazioni, o meglio le condivisioni dei *post*, erano coperte dalla causa di non punibilità, espressa all'articolo 68 della Costituzione; secondariamente, senza subordine alcuno e dalla superiore eccezione, quell'ufficio ritiene la non sussistenza del reato ipotizzato e che la mia condotta invece è più realisticamente espressione del diritto di critica: «Nel caso in esame, i parametri guida risultano rispettati, con la conseguenza che non può ritenersi diffamatorio il contenuto di quanto pubblicato e condiviso sui *post*. A tale proposito, si evidenzia come le espressioni utilizzate risultino prive di espressioni offensive, non risolvendosi in alcun modo in un attacco personale e gratuito». Proprio nel solco di quanto finora delineato, la mia condotta si inquadra nel diritto di critica. Per queste argomentazioni e considerato che non sarebbe fondamentale e sostenibile l'accusa in giudizio e quindi pervenire con certezza a una sentenza di condanna, proprio per l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato, il sostituto procuratore Francesco Caporale e il pubblico ministero Erminio Amelio hanno chiesto al giudice delle indagini preliminari l'archiviazione del procedimento, stante l'infondatezza del reato.

la finalità postuma della gogna era di impedirmi di presiedere la Commissione d'inchiesta sulle banche, per il terrore che avrei potuto scoperchiare sepolcri imbiancati: da Banca Etruria al buco nero di MPS, che ha bruciato 60 miliardi di euro. *(Applausi)*. Nell'Italia tra i primi posti per corruzione e tra gli ultimi per libertà di stampa, le due facce della stessa medaglia, mentre vi furono oltre mille articoli sull'accusa di odio razziale e centinaia di *talk show* in televisione, l'archiviazione ha avuto tre miseri articoli sui media.

Fosse anche l'ultima azione della mia vita, li citerò in giudizio tutti a rispondere di quelle calunnie: giornalisti, politici e commentatori,

Signor Presidente, voglio portare all'attenzione di quest'Assemblea e dei competenti organi la grave situazione che riguarda l'emergenza idrica nella provincia di Agrigento. una seria problematica, che ormai va avanti da molti anni e che riguarda la vita quotidiana di decine di migliaia di persone, in un'area peraltro cronicamente carente di infrastrutture e con un'economia fragile; il tutto, aggravato dall'emergenza Covid-19. Negli ultimi mesi, questa situazione è ulteriormente peggiorata dopo il dissesto finanziario e il conseguente commissariamento della società Girgenti Acque SpA, alla quale era affidata la gestione del servizio idrico.

di un'interruzione dell'erogazione dell'acqua. Oltre alla questione idrica, c'è anche il gravissimo problema occupazionale, con 300 lavoratori della Girgenti Acque che rischiano di trovarsi senza lavoro, con disastrose ripercussioni sulla vita delle loro famiglie. Il commissario prefettizio della società Girgenti Acque è stato chiarissimo: se non si interviene subito, ci sarà la sostanziale impossibilità di far fronte agli obblighi economici, anche minimi, nei confronti dei fornitori, rendendo così impossibile il funzionamento del sistema. Questa è una situazione insostenibile. È inaccettabile, infatti, che un certo cronico lassismo dei competenti organi possa avere tali conseguenze su centinaia di lavoratori e su migliaia di cittadini, che potrebbero trovarsi senz'acqua addirittura nel mese più caldo dell'anno, con gravissime ripercussioni non solo sulla vita quotidiana, ma anche sulla stessa salute, già fortemente minata dalla pandemia, che peraltro è in forte ripresa. Con questo mio intervento rivolgo quindi un appello pubblico alla Regione Sicilia, affinché prenda in mano la situazione, assumendo provvedimenti urgenti e risolutivi. Chiedo altresì che tali interventi siano improntati alla massima trasparenza, per evitare che si ripetano gli episodi di opacità fin qui accaduti. L'intera popolazione agrigentina attende con grande preoccupazione i prossimi accadimenti. Decine di città sono coinvolte. È il momento di interventi urgenti. Per quanto mi riguarda, continuerò a occuparmi con forza del mio territorio, senza polemiche inutili, ma guardando soltanto alla concretezza delle azioni e al benessere della nostra cittadinanza.

in queste ultime tre settimane ho fatto un breve *tour* in alcune carceri. Voglio raccontare in quest'Aula ciò che mi è occorso venerdì 23 luglio, durante la visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Ritengo doveroso infatti che Esecutivo e Parlamento abbiano un confronto su una problematica così delicata e, allo stesso tempo, così spigolosa come quella che attiene alla situazione carceraria del nostro Paese.

nonostante la recente visita in quel luogo da parte della ministra Cartabia e del presidente del Consiglio Draghi. Ribadisco trattarsi di un fatto di imbarazzante gravità: vengo accolta e accompagnata da una persona che non si presenta, in abbigliamento sportivo, facendo presupporre di essere un poliziotto in borghese, il quale mi accompagna prima dalla direttrice, poi mi fa da cicerone nel reparto delle detenute, dando indicazione alle commissarie di aprire l'aula della sartoria e mostrandomi lì le mascherine contro la violenza sulle donne, tema che a noi sta molto a cuore; continua poi a dare indicazioni alla commissaria

Immaginate il mio grande stupore nell'apprendere questa notizia, dal momento che ero lì senza autista, come mia consuetudine. Leggo il nome del presunto autista, tale Armando Schiavo. Chiedo a gran voce chi sia costui: all'ennesima mia richiesta,

del personale, in cui risulta che l'uomo, il presunto autista, Armando Schiavo, è autorizzato a entrare nel carcere per finalità rieducative e frequentare esclusivamente il laboratorio di pasticceria suo interno, che opera solo nella giornata di martedì. Il provvedimento è stato emesso dopo la valutazione da parte del DAP di atti dell'istituto penitenziario e della magistratura di sorveglianza. Il DAP sta valutando attualmente la scelta della dirigente, Elisabetta Palmieri, che verrà sostituita fino alla nomina del nuovo direttore.

i Capigruppo hanno convenuto che il testo del maxiemendamento, non appena pervenuto, anche a seduta sospesa, sarà immediatamente trasmesso alla Commissione bilancio, che è autorizzata a convocarsi per esprimere il parere sui profili di copertura finanziaria. La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 22,30.

alle ore 22,31)*. Informo che il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo del decreto-legge all'ordine del giorno, che è stato trasmesso alla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, per i profili di copertura finanziaria. In attesa del parere della 5a Commissione, sospendo la seduta.

Informo che la 5a Commissione permanente ha reso il parere sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.9000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo del decreto-legge. Invito il senatore Segretario a dare lettura di tale parere. Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni

relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 3, comma 4, lettera *a)*, dopo le parole: "cinquanta per cento dei posti", siano inserite le seguenti: "calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati,"; all'articolo 3, comma 4, lettera *b)*, dopo le parole: "anche da membri esterni", siano inserite le seguenti: "senza maggiori oneri per la finanza pubblica", e dopo le parole: "non superiore a tre anni.", sia aggiunto il seguente periodo: "L'applicazione della disposizione di cui al presente comma non deve determinare posizioni sovrannumerarie."; sia soppresso il comma 10-*ter* dell'articolo 3; - all'articolo 17-*terdecies*, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190". In conformità all'articolo 161, comma 3-*ter*, del Regolamento, la Presidenza ha valutato il testo dell'emendamento, ai sensi degli articoli 8 e 97 del Regolamento. Prende atto delle condizioni poste dalla Commissione bilancio relativamente all'articolo 3, comma 10-*ter*, e provvede allo stralcio dell'articolo 17-*terdecies* per estraneità di materia. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà.

Probabilmente c'è una qualche estraneità della materia, ma credo che il Parlamento italiano meriti rispetto. *(Applausi)*. Pertanto, è giusto che prendiamo atto della sua decisione, ma domani presenteremo un disegno di legge perché si faccia immediatamente la proroga di quei tribunali.

Caliendo, mi preme fare una precisazione, perché è nota a tutta quest'Assemblea la difesa che ho sempre fatto, dall'inizio di questo mandato, della

tutto l'*iter* procedimentale di questo difficile provvedimento,

e sicuramente vi avranno reso edotti di tutto quello che oggi pomeriggio è stato discusso in Conferenza dei Capigruppo e di come sono andate le cose).

Mi meraviglio, perché lei di solito non ha di queste espressioni.

non si può nemmeno dire che ce lo chiede l'Europa, perché ci chiede l'esatto contrario, ossia la giustizia di prossimità. C'è un'infinità di motivazioni per tenere aperti quei tribunali, ma non voglio fare un discorso territoriale, bensì uno generale. Il Parlamento, signor Presidente, ha espresso un emendamento, con grande fatica, in modo unanime.

Presidente, con tutto il rispetto che posso avere della Presidenza, essendo stato anche un esponente di Governo, mi permetta di dire che lei non sta svolgendo equamente il suo ruolo e non difende nessuno dei parlamentari presenti in quest'Aula.

secondo un rigore logico, il fatto che lei abbia dichiarato inammissibile l'emendamento è insindacabile, ma, secondo lo stesso criterio logico, non è detto che ciò che è insindacabile sia giusto.

della democrazia. Se maggioranza e opposizione compiono uno sforzo, vuol dire che questo ha un senso. *(Applausi)*. Allora, nel metodo e nel nel merito, penso - perché me lo hanno insegnato quando andavo a scuola - che il Parlamento sia sovrano. Signor Presidente,

tra un giovedì e un venerdì di fine luglio, una Commissione che si sforza di trovare delle coperture? Vorrei sapere che gioco è questo come si chiama: è il gioco dell'oca? Che cos'è? Qui non siamo stati eletti per giocare e non veniamo a quest'ora per giocare. Trovo che quello che si sta verificando stanotte - e mi auguro che al di fuori dell'Aula

signor Presidente, rispetto lei, come persona, e la sua figura, ma non posso non dire, come Fratelli d'Italia, che tutto questo è surreale, offensivo e direi anche umiliante e, quando si umilia un'Assemblea parlamentare, si viene meno ad alcuni principi di fondo. Non veniamo qui per lavorare a vuoto ed essere presi in giro. Senatrice Rauti, lei ha fatto riferimento a un concetto di democrazia, e ci mancherebbe altro che non venisse rispettato il principio democratico proprio qua dentro, in un Senato che è la culla della democrazia.

che va rispettata sempre e comunque, dentro un perimetro di diritto. C'è anche una volontà politica che non entra nel perimetro del diritto, perché la valutazione di estraneità

le ragioni che spingono a questa protesta. Lo capisco esattamente. Sto dicendo semplicemente che, come ha detto prima il senatore Caliendo, questa volontà politica si può esprimere in un disegno di legge concorde, che può passare con un articolo in sede deliberante;

di non esercitare più pienamente il nostro ruolo, nel senso che le nostre prerogative vengono regolarmente calpestate. Signor Presidente, ha fatto bene a richiamare le regole: è vero, la democrazia è fatta

Non possono essere applicate in modo unilaterale solo in alcuni casi. *(Applausi)*. Questo è il problema fondamentale che abbiamo, ha capito?

Siamo qui dalla mattina alla sera solo e unicamente a convertire decreti-legge, senza neanche poterli leggere, com'è successo ieri. Questo è quella a cui siamo ridotti.

come l'abbiamo detto altre volte - che si continui a calpestare così la democrazia parlamentare. Non è più possibile. C'è un problema molto serio in questo Paese.

autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento che recepisce integralmente le proposte emendative approvate dalle Commissioni riunite e interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2272, di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nel testo dichiarato proponibile dalla Presidenza, accogliendo altresì le condizioni formulate nel parere della Commissione bilancio. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo

come opposizione, abbiamo collaborato pienamente. Ringrazio i relatori, i senatori Caliendo e Valente, e la sottosegretaria Bini. Abbiamo portato numerosi emendamenti e diversi sono stati approvati. Avremmo dovuto continuare questo lavoro in Aula, perché quello in Commissione è finito ieri alle ore 20. Sono passate ventotto ore, avremmo potuto lavorare da questa mattina fino ad ora

un provvedimento non secondario nell'ambito di un disegno di legge che reca misure urgenti per l'efficientamento della pubblica amministrazione e per l'efficienza della giustizia. giustizia. Avremmo voluto svolgere un dibattito vero anche in Aula per migliorare ulteriormente un provvedimento in cui abbiamo riscontrato diversi aspetti positivi, per questo abbiamo collaborato a migliorarlo, così come delle carenze. I colleghi di Fratelli d'Italia che sono intervenuti, i senatori Iannone, Zaffini e Balboni, hanno portato diversi contributi importanti riguardanti due questioni in particolare: quella della giustizia e quella della sanità. È curioso che, nell'ambito di provvedimenti che vengono a seguito della pandemia, la sanità abbia una parte una parte molto marginale, anche se ha una grossa carenza di personale, non solo per la pandemia, ma anche per il gran numero di pensionamenti e una carenza che già c'era in precedenza; in più, siamo in una situazione particolare, per cui ci sarebbe stata la necessità di valorizzare davvero questo settore. Quanto al comparto della magistratura, c'è stata solo quest'attenzione all'ufficio del processo, con una serie di problemi che il senatore Balboni

nello smaltimento del grande arretrato che c'è nella giustizia. L'emendamento non è stato approvato. Non si è fatto nulla sulla magistratura onoraria, onoraria, che lodevolmente porta avanti una parte importantissima del lavoro della giustizia, e anzi, nonostante l'impegno del ministro Cartabia di portare una proposta entro il 30 giugno su questo importante settore, ci si è dovuti ridurre a un emendamento, presentato all'ultimo momento, che proroga ancora la situazione attuale, senza risolvere il problema, né ottemperare alle richieste dell'Unione europea, che chiede che questa categoria goda finalmente di una decente e giusta collocazione e delle tutele opportune. La pubblica amministrazione è importantissima nel nostro Paese (e non solo da noi, naturalmente) e dobbiamo valorizzare questo settore importantissimo, che non può essere visto solo come un costo da tagliare, ma come una grande risorsa su cui effettivamente si spende una parte importante del bilancio del nostro Paese e dunque dev'essere valorizzata;

bravissimi ed encomiabili dipendenti pubblici di tutti i livelli, che svolgono un lavoro importantissimo. Bisogna fare in modo che questo grande apparato sia ancora di più al servizio dei cittadini, che sia lì per risolvere i problemi, come tantissimi pubblici dipendenti e dirigenti fanno, e che non appaia mai come quello che invece cerca di frenare bloccare le iniziative dei privati. Ci vuole veramente una sinergia di questo settore con l'intero Paese e con l'intero apparato produttivo

nelle Commissioni riunite. Credo che tutti i senatori abbiano il diritto di intervenire su argomenti estremamente importanti. Il tempo c'era tutto, ma evidentemente si è voluto tarpare

insindacabile parere da quello che ha già inserito il Governo, non si può fare nulla. Di conseguenza, la funzione legislativa che la Costituzione assegna senza ombra di dubbio al Parlamento viene spostata altrove, con mancanza di trasparenza, per cui non c'è mai nessuno che si assuma veramente la responsabilità sulle singole parti di provvedimenti molto ampi,

voteremo ovviamente contro la fiducia, pur esprimendo apprezzamento per molte parti di questo provvedimento, che vanno in direzione della valorizzazione della pubblica amministrazione.

concorsuali e in tutti i tipi di assunzione. Lo Stato non deve in nessun modo far passare il messaggio che si entra nella pubblica amministrazione per ragioni diverse dal merito e su questo ci saremo sempre. Votiamo contro la fiducia ma, quando si tratta di lavorare per gli interessi degli italiani, ci siamo sempre. Signor Presidente, considerate le circostanze, il mio sarà un intervento molto breve. Ci troviamo in un momento particolare della storia del nostro Paese e dell'Europa, abbiamo bisogno di riforme profonde della pubblica amministrazione e della giustizia, sappiamo di essere nel dovere più pieno di sfruttare le risorse che il PNRR mette a disposizione del nostro Paese, a fronte della certezza di interventi che siano in grado di rinnovare e potenziare la nostra pubblica amministrazione e il nostro servizio della giustizia. Il provvedimento va in questa direzione, ha attraversato il processo di conversione in Parlamento, con un lavoro importante e molto difficile sotto tutti i punti di vista, che si è svolto nella Commissione in un clima collaborativo tra i vari livelli delle istituzioni che si sono trovati a interagire e anche tra maggioranza e opposizione. Credo siano stati apportati miglioramenti equilibrati e si sono dovute anche fare scelte difficili delle quali è stato necessario farsi carico. Ritengo che sia importante aver inserito elementi di accelerazione e di sveltimento nelle procedure di reclutamento e, per quanto riguarda il settore della giustizia, c'è la grande scommessa della costituzione dell'ufficio per il processo con tante assunzioni. Bisogna non soltanto assumere tanto, ma anche assumere le figure giuste e inserirle nel sistema i miglioramenti che sono stati apportati in Parlamento, si è avuto riguardo per esigenze poste al Parlamento dagli enti locali, dando ad essi una risposta a mio avviso equilibrata, attraverso emendamenti presentati da tutti i Gruppi. Mi pare che in un giorno che registra, a livello nazionale, un passo avanti importante, anche all'interno della maggioranza, su una riforma cruciale come quella della giustizia, il Senato approvi un provvedimento che va nella direzione corretta. Per questo il Partito Democratico voterà a favore del provvedimento

ma ovviamente speriamo che l'immissione nella pubblica amministrazione e negli enti territoriali di forze giovani e iperqualificate possa essere di per sé Grazie a tutti

Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, siamo al termine di due giorni di lavoro impegnativo

Mi interessa in questa sede, signora Presidente, evidenziare ancora una volta una sorta di invasione di campo da parte degli organi governativi e della burocrazia ministeriale nei confronti del Parlamento. Non è la prima volta. Credo di essere stato il primo a sollevare questo problema in uno dei provvedimenti approvati passato, ma credo che oggi abbiamo raggiunto il culmine di questa interferenza. Lei ha esercitato una sua prerogativa, e su questo nessuno ha da dire nulla, però sapevamo che su quel famoso emendamento che prorogava soltanto di due anni alcuni tribunali minori dell'Abruzzo vi era una ferma opposizione da parte del Ministero della giustizia, una opposizione degna di miglior causa, come per esempio quella di mantenere ferma una riforma sulla giustizia che, leggendo i giornali di questa mattina, sembra sia stata annacquata. Quindi, quella fermezza che il Ministero della giustizia ha tenuto su questo emendamento, ben avrebbe potuto essere esplicitata nel mantenere fermi e saldi alcuni principi della riforma della giustizia, ma questo è un discorso che prima o poi dovremmo affrontare.

con l'emendamento sull'Abruzzo, che il Parlamento non è disposto a farsi dettare le regole dal Governo, né dai burocrati *(Applausi)*, perché in questo Paese il potere legislativo appartiene soltanto al Parlamento e a nessun altro, né al Governo, né ai burocrati ministeriali.

Puntiamo sulla meritocrazia e grazie all'acume e all'intuizione del Ministro per la pubblica amministrazione, puntiamo su procedure più snelle e più rapide per il reclutamento, che fino ad ora avevano imbrigliato le pubbliche amministrazioni. Ci auguriamo che questa ventata di novità possa essere utile anche ad un salto culturale all'interno della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda la giustizia,

espletato la sua attività e dovrà tornare in gran parte a casa. Forse sarebbe stato meglio assumere o creare delle sezioni stralcio, come è stato fatto negli anni passati, per azzerare l'arretrato,

creare un'Assemblea costituente, visto che né le bicamerali, né le riforme fatte dalle varie maggioranze costituzionali hanno avuto fortuna. Forse dovremmo convincerci che l'unica strada per modernizzare il nostro Paese è quella di creare una Assemblea costituente. Quindi, con queste considerazioni, esprimo il voto favorevole del Gruppo al provvedimento

Anche io ringrazio tutti coloro che hanno lavorato al provvedimento in esame: i relatori, il Governo, i membri delle Commissioni e in modo particolare gli Uffici, che ci hanno assistito.

Vorrei ricordare che abbiamo introdotto emendamenti che valorizzano il portale del reclutamento, che ora diventa portale unico del reclutamento e della mobilità nella pubblica amministrazione. Ciò serve a dare maggiore trasparenza, prevedendo che i bandi per il reclutamento del personale siano pubblicati come documenti in formato aperto e organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo, in modo tale che tutte le procedure di reclutamento - e in particolar modo quelle per la mobilità del personale degli uffici pubblici - diventino più trasparenti. Infatti, fino ad oggi, come ammesso anche dal ministro Brunetta, la mobilità nella pubblica amministrazione è una procedura opaca.

condiviso da più forze politiche, che prevede l'assunzione di 184 nuove unità di personale a favore dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Si tratta di un importante tassello che va ad aggiungersi a quanto già previsto con le assunzioni previste dal PNRR e che è utile a rafforzare la tutela e la sicurezza dei lavoratori in una stagione in cui i morti sul lavoro sono tre ogni giorno. per contrastare il lavoro sommerso e irregolare, una piaga che va combattuta con determinazione e azioni concrete, anche per garantire il rispetto delle regole di mercato e, quindi, lo sviluppo di un'imprenditoria sana. In generale che cosa vogliamo con queste misure e risorse approvate? Quello che vogliamo è una pubblica amministrazione rinnovata, in grado di ascoltare le richieste dei cittadini e delle imprese, capace di dare risposte e servizi in maniera efficace ed efficiente. Questo rinnovamento si deve basare su alcuni assi importanti. Il primo è la trasformazione digitale: una pubblica amministrazione digitalizzata e sburocratizzata è in grado di interagire più rapidamente con le persone e le aziende. Sappiamo che nella pubblica amministrazione i laureati sono cresciuti, ma negli ultimi dieci anni vediamo che

che, attraverso il loro lavoro, sappiano orientare le decisioni politiche. Le competenze informatiche, anche a livello dirigenziale, sono fondamentali per non fallire ancora nella trasformazione digitale. Come MoVimento 5 Stelle ci batteremo sempre per un sistema di reclutamento e progressione aperto, equo e meritocratico, che oggi ancora trova troppi ostacoli nella politica e nelle amministrazioni. Vogliamo una pubblica amministrazione specchiata, che sia veramente capace di mettere al centro il cittadino e i suoi bisogni. Per questi motivi, anche per questa volta, rinnoviamo la fiducia al Governo.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

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021,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

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di